ieri il Senato ha avuto al suo interno un confronto importante, responsabile e significativo che non ha trovato una corretta comunicazione esterna. Mi riferisco in particolare ai servizi del TG1 che si sono limitati a comunicare l'avvenuta approvazione del provvedimento così come licenziato dalla Camera dei deputati. Questo è un elemento di disinformazione che non rende onore al dibattito che si è svolto in Senato. Desideravo segnalarlo perché in termini di comunicazione istituzionale si dia alla pubblica opinione una corretta informazione del lavoro di questo

*relatore*. Signor Presidente, in primo luogo è utile un esame delle soluzioni adottate o non adottate sulle questioni che in questa stessa sede sollevammo l'anno scorso. Nel condurre questo confronto si impone un *caveat*. L'anno scorso discutemmo il bilancio preventivo 2006 e il consuntivo 2004 nell'ottobre 2006, quasi alla fine dell'anno. Le soluzioni adottate vanno quindi commisurate - oggi siamo ad aprile - al brevissimo lasso di tempo intercorso tra il voto di approvazione di quel bilancio e l'odierna seduta, in tutto cinque mesi. mesi. Dobbiamo avere pertanto questa avvertenza. Inizio dalle questioni che sono state risolte o almeno, a mio giudizio, positivamente affrontate. I documenti di bilancio di previsione al nostro esame sono stati predisposti in febbraio e sono in fase di approvazione all'inizio di aprile, mentre sono stati predisposti e possono essere esaminati e approvati dall'Assemblea il rendiconto 2005 registriamo alcuna novità perché abbiamo sempre avuto una distanza di due anni in termini di approvazione del rendiconto) e il rendiconto 2006 (qui invece la novità c'è perché per la prima volta nell'anno immediatamente successivo discutiamo il rendiconto); dunque, c'è un passo avanti che consente di mettere su basi più certe la decisione circa le scelte allocative nel bilancio di previsione, perché consente a queste scelte di radicarsi

L'anno scorso sollevammo con forza il tema che, con un termine orribile ma che rende l'idea, chiamammo l'intercameralità di alcuni servizi fondamentali. Se è persino ovvio che - a Costituzione vigente e cioè a sistema di bicameralismo perfetto - ciascuna Camera si doti autonomamente dei servizi essenziali allo svolgimento della sua specifica attività, è assai meno comprensibile - e in ogni caso fonte di inefficienze e di duplicazioni di spesa, a mio giudizio inaccettabili - che ciascuna Camera operi in perfetta autonomia dall'altra laddove si tratta di servizi e attività che dovrebbero essere - e come tali sono naturalmente concepiti nel Paese - propri del Parlamento nel suo complesso e non di ciascuna Camera autonomamente.

ma una sede unitaria dove la banca dati è unica o quasi e le politiche di acquisto sono coordinate. Con questo esempio abbiamo dimostrato che si può ottenere risultato con questa iniziativa. In un campo immediatamente contiguo, quello degli archivi storici di Camera e Senato, si potrebbe - e secondo me si dovrebbe - fare esattamente la stessa cosa. Qui però le sedi fisiche sono ubicate in modo tale che non basta, com'è accaduto per la biblioteca, aprire una porta per mettere le basi del processo di unificazione. Signor Signor Presidente, soprattutto credo che lei, in accordo con il Presidente della Camera, dovrebbe porsi il problema di ridurre i costi migliorando il servizio. Se la struttura è una, le attività di direzione possono essere unificate e il personale, almeno in parte, ridotto. Pur senza puntare all'unificazione, un forte e ben organizzato coordinamento appare possibile e, a mio giudizio, auspicabile anche per i due Servizi studi; mentre un processo di vera integrazione si può e si deve realizzare per il Servizio internazionale, come ha sottolineato in particolare il Presidente della Commissione affari esteri del Senato nella riunione dei Presidenti che ha preceduto e preparato questa relazione. Il Servizio del bilancio, inteso in particolare come sede di costante monitoraggio dei conti pubblici e di corretta valutazione degli effetti economici e sociali delle scelte allocative e di garanzia della trasparenza dei conti pubblici, può essere unificato attraverso la creazione del Servizio di bilancio del Parlamento italiano, ferma restando l'esigenza di mantenere al suo interno attività dedicate all'esame tecnico delle coperture finanziarie della nuova legislazione di spesa e di entrata in riferimento ai lavori di ciascuna Camera. Se inserisco questo tema in questa parte della relazione - quella che esamina i problemi affrontati, se non totalmente risolti - non è ovviamente perché l'obiettivo proposto sia stato conseguito, ma perché si sono compiuti e si stanno compiendo passi importanti nella direzione indicata, cosa della quale ringrazio naturalmente il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei senatori Questori. In primo luogo, si stanno utilizzando le risorse permanenti a ciò dedicate dalla legge finanziaria 2007: il Consiglio di Presidenza ha infatti bandito - nella relazione scritta avevo dovuto scrivere ancora «sta infatti bandendo» perché il bando è stato pubblicato ieri - il concorso per l'assunzione permanente di un numero ristretto di unità di personale dotato dell'elevata e specialissima qualificazione necessaria. In secondo luogo, è stata individuata una figura che dovrebbe svolgere il lavoro di analisi degli andamenti di finanza pubblica in Senato operando in coordinamento con l'analogo Servizio della Camera dei deputati. In terzo luogo, il Consiglio di Presidenza ha deciso, nelle more dello svolgimento del concorso cui abbiamo accennato, di ricorrere al contributo temporaneo di risorse già operanti in altre istituzioni o istituti di ricerca. Dato il tempo trascorso da quando abbiamo sollevato formalmente il problema - cioè cinque mesi - e avanzato la proposta, non mi sembra che il cammino percorso possa essere considerato irrilevante. Ad accompagnare gli sforzi del Consiglio di Presidenza può e deve ora intervenire la formazione, in seno alla Commissione bilancio, di un apposito Sottocomitato per la trasparenza e il monitoraggio dei conti pubblici che, lavorando di concerto con quello analogo che verrà costituito presso l'analoga Commissione della Camera dei deputati, fornisca il necessario supporto politico, rigorosamente *bipartisan*, all'avvio di questa nuova, per il Parlamento, attività di monitoraggio e controllo. La nascita di questo Sottocomitato presso la Commissione bilancio non deve trarre in inganno i Presidenti e i senatori delle altre Commissioni: l'attività del futuro auspicabile Servizio del bilancio del Parlamento italiano risulterà indispensabile per tutte le Commissioni, anche per la sua crescente capacità di mettere in relazione risorse impiegate e *performance*, sottoponendo a verifica le previsioni originarie, cioè quelle effettuate al momento della prima approvazione della legislazione di spesa o di entrata. Nella relazione e nel confronto sul bilancio 2007 ponemmo infine l'accento sul tema dell'allocazione delle diverse attività nelle diverse sedi a disposizione del Senato: le attività di autoamministrazione più lontane, dicemmo, e le attività di *core business* del Senato, cioè legislazione e sindacato sul Governo, nelle sedi più centrali. Sento l'esigenza di un rendiconto più puntuale, a questo proposito, del lavoro svolto, ma - sempre assumendo a riferimento i cinque mesi intercorsi - mi sembra che siano stati compiuti passi nella direzione giusta. Numerosi Presidenti di Commissione hanno fatto tuttavia osservare, signor Presidente, anche quest'anno, che gli spazi fisici messi a disposizione per la specifica attività di Commissione permangono deficitari per quantità e qualità, mentre la programmazione dei lavori dell'Aula rende incerti i calendari di attività delle Commissioni stesse, così accentuando il già significativo disagio derivante dalla non eccelsa qualità delle sedi. Venendo ora ai temi su cui non si è potuto (oppure, in piena legittimità, intendiamoci bene, voluto) intervenire, riprendo brevemente il tema della natura del nostro bilancio: soltanto di cassa, come è, o anche di competenza, come qualcuno - tra i quali il sottoscritto Abbiamo già dovuto prendere atto, lo scorso anno, della scelta del Regolamento di amministrazione e contabilità di non adottare il criterio della competenza. Capisco, anche se fatico - lo dico sinceramente - ad adeguarmi. Gli allegati previsti dal comma 6 dell'articolo 2 del Regolamento sono certamente utili e appaiono in grado di dare conto, almeno in parte, degli effetti, nei periodi successivi a quelli in esame, delle obbligazioni assunte. È tuttavia la stessa relazione dei senatori Questori al nostro esame a dare conto delle difficoltà implicite nel metodo prescelto, cioè quello della cassa, sia laddove raccomanda una riforma del regolamento contabile per dare carattere «strutturale» al trasferimento di quote dell'avanzo al secondo anno successivo a quello di riferimento (quale migliore dimostrazione di una specie di desiderio di un bilancio di competenza di questa frase), sia laddove non offre adeguate informazioni sulle prevedibili evoluzioni della futura spesa previdenziale del Senato, che è una componente fondamentale del bilancio. Bene, quindi, la raccomandazione sulla riforma del Regolamento, ma insistiamo: perché non elaborare, per grandi aggregati di spesa e di entrata e a meri fini conoscitivi almeno, uno schema di bilancio di competenza che dia il senso del carattere pluriennale degli impegni che vengono assunti? Lo scorso anno, signor Presidente, segnalammo l'anomalia e i rischi insiti nella mancata definizione del trattamento previdenziale dei dipendenti del Senato assunti dopo il 1998. Anche se la nostra sollecitazione non è caduta nel vuoto, anzi so che il Consiglio di Presidenza sta procedendo nella direzione che l'anno scorso ci permettemmo di indicare, non è tuttavia ancora questo confronto entrato in una fase risolutiva entrato in una fase risolutiva per l'adozione di un nuovo sistema previdenziale che introduca per i dipendenti certezza dei diritti e per il Senato certezza dei costi. Non ci resta che sollecitare ulteriormente l'accelerazione di questo confronto, ribadendo ciò che - in termini di metodo - facemmo notare lo scorso anno: se il salto di qualità nel sistema previdenziale pubblico italiano è stato ed è rappresentato dall'adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, appare ragionevole e, soprattutto, politicamente sostenibile, nel rapporto col Paese - una soluzione che, a regime, presenti caratteri analoghi, cambiato tutto quello che c'è da cambiare. Ferma restando - come per il cosiddetto sistema Dini - una fase di transizione al regime di calcolo contributivo che mantenga il metodo di calcolo retributivo per il personale più anziano e adotti il metodo del cosiddetto *pro rata temporis* (gli esperti di previdenza sanno a che cosa mi riferisco) per gli assunti più di recente. Analogamente - e in coerenza col confronto in atto nel Paese sullo stesso tema - dovrebbe essere affrontata l'ineludibile questione dell'età di pensionamento per il personale che mantiene il calcolo retributivo, perché per quello che avesse il calcolo contributivo il problema, come è noto, non si porrebbe. A proposito di chi mantiene il calcolo retributivo, si pone, com'è noto, il problema del salto in aumento: tutto in un'unica soluzione (nel gergo politichese lo scalone), oppure incrementi progressivi (nel gergo politichese gli scalini)? Con lo stesso spirito, dovranno essere affrontati i problemi posti dalle aliquote contributive, che, se appaiono vicine e anche superiori a quelle in atto nel sistema pubblico per la quota a carico del lavoratore, appaiono implicitamente (dico «implicitamente» perché il loro importo non è formalmente determinato, nemmeno in via figurativa) molto distanti, per difetto, sia da quelle di computo sia da quelle di equilibrio, determinando così le basi strutturali per uno squilibrio strutturale del sistema. Presidente, non appaiono ben definite e motivate, inoltre, le ragioni che inducono a rimpinguare i fondi di riserva (si veda pagina 19 della relazione dei senatori Questori), tanto più che l'aumento nel complesso, tra parte corrente e parte capitale, si presenta molto forte rispetto al preventivo (+17,65 per cento) e fortissimo in rapporto all'assestamento. Non si nega che da queste decisioni relative ai fondi di riserva derivi (per quanto non risulti immediatamente intuitivo) maggiore trasparenza, perché la flessibilità del bilancio da questo lato - dal lato dei fondi di riserva viene compensata dalla puntualità delle previsioni sulle altre voci di spesa e di entrata. Ma resta il fatto che ci sia bisogno di una più analitica indicazione delle ragioni che determinano le scelte relative all'impinguamento così rilevante dei fondi di riserva. Con riferimento alla necessità di un riorientamento delle risorse a favore del cosiddetto *core business* (legislazione e sindacato sul Governo) rispetto ad attività non direttamente connesse a questo fulcro, vanno certamente apprezzate prime scelte di riequilibrio, che mostrano l'evoluzione della spesa nel secondo comparto. Anche al fine di meglio documentare e controllare, da parte dell'Assemblea, il costante progresso in questo campo, appare certamente utile un'ulteriore operazione di accorpamento o selezione delle aggregazioni di bilancio per aree omogenee, al fine di far emergere che l'area di attività di documentazione (si è già detto, a titolo di esempio, del Servizio del bilancio) subisce, nell'ambito della ristrutturazione già in corso, un progressivo rafforzamento (risorse finanziarie, umane e non solo) a scapito di quelle di autoamministrazione della struttura, che devono scendere a livelli percentuali di spesa decisamente inferiori, a mio giudizio, rispetto agli attuali. Allo stesso modo, la particolare attività dell'istituzione sembra reclamare la determinazione di una specifica area di intervento in tema di formazione continua del personale (non ho bisogno di spiegare perché necessitiamo di un continuo miglioramento delle *performance* qualitative del personale di un'istituzione autorevole come il Senato). Quanto alla regolazione delle acquisizioni di beni e servizi da soggetti esterni o alle esternalizzazioni di attività precedentemente svolte «in casa», si possono avanzare due suggerimenti, tra di loro strettamente connessi: da un lato, il ricorso alla trattativa privata con produttori esterni appare da sconsigliare - malgrado presenti evidenti vantaggi di celerità - quando si applichi a singole componenti di un intervento unitario o di maggiori dimensioni. l'esperienza di questi anni sembra suggerire gare per l'acquisizione di «servizi globali», i cui prestatori sono in grado di realizzare rilevanti economie di scala, per un migliore processo di ottimizzazione dei costi. Nella riunione dei Presidenti di Commissione che ha preceduto questa seduta, i senatori Questori hanno dato conto delle iniziative del Collegio in questo senso, incontrando unanime apprezzamento. Con riferimento alla politica del personale (questo è un punto di particolare rilievo, signor Presidente, che vorrei sottolineare per l'attenzione sua, dei senatori Questori e di tutti i senatori),

(sottolineo «più propriamente») «ricondotto al parametro dei dipendenti presenti in pianta organica», piuttosto che al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2006. Signor Presidente, devo prenderne atto, ma debbo segnalare che tale orientamento si pone in aperto contrasto con quello costantemente praticato dalla Commissione bilancio del Senato (in questa come nelle precedenti legislature, in verità), che ha sempre preteso dal Governo - in sede di esame della legislazione per i profili di copertura finanziaria - il riferimento agli organici di fatto, non a quelli di diritto, per la ragione ovvia che, se l'obiettivo è quello del contenimento della spesa, esso potrà dirsi conseguito solo se diminuisce il numero delle persone effettivamente in servizio, non se diminuisce rispetto ad un numero di dipendenti scritto sulla carta che non esiste nella realtà. infatti notare che la pianta organica prevede un numero di dipendenti decisamente superiore a quelli ancora attualmente in servizio, che pure sono già aumentati nel quinquennio appena trascorso di quasi il 30 per cento in termini di unità. Quanto alla prevista evoluzione delle retribuzioni, la relazione dei senatori Questori segnala una sensibile contrazione degli aumenti rispetto a quanto previsto nel

che il ritmo di crescita si manterrebbe ben al di sopra del tasso di inflazione programmata, come è avvenuto negli anni scorsi, con effetti cumulati che sono davvero impressionanti se si guarda all'evoluzione degli ultimi dieci anni. Infine, qualche valutazione sul tema dell'equilibrio finanziario del sistema degli assegni vitalizi dei senatori cessati dal mandato. I prossimi mesi, colleghi senatori, saranno caratterizzati da un vasto confronto nel Paese sul sistema previdenziale pubblico. Il Governo e le parti sociali ne stanno discutendo proprio in queste ore, con l'obiettivo di garantire una migliore sostenibilità sociale e finanziaria del sistema. Signor Presidente, gli assegni vitalizi degli ex parlamentari non sono, tecnicamente, «pensioni», ma per ogni cittadino italiano il vitalizio il vitalizio è la «pensione» dei parlamentari. È dunque decisivo - per la credibilità delle istituzioni e la legittimazione di ognuno di noi ad essere protagonista del discorso pubblico in tema di previdenza

sottodeterminate rispetto al livello delle prestazioni, con uno squilibrio impressionante e a mio giudizio economicamente insostenibile; alle regole del riscatto delle mancate contribuzioni, troppo favorevoli;

ma non c'è dubbio che su questo punto resta per il pregresso una situazione difficilmente sostenibile. L'intervento riformatore realizzato nella XIII legislatura ha certamente un suo rilievo, specie per il drastico innalzamento dell'età anagrafica di accesso alle prestazioni. Così come ha un effetto positivo la scelta di aver posto a carico dei senatori lavoratori dipendenti iscritti ai sistemi previdenziali pubblici il pagamento di una quota dei contributi

la piena compatibilità politica del sistema dei vitalizi degli ex parlamentari con i pilastri portanti del sistema previdenziale pubblico e la sua migliore sostenibilità finanziaria. Una sostenibilità che i dati di bilancio (contributi *versus* prestazioni) dimostrano precaria (ed è un eufemismo), anche a causa dell'assenza di una qualche forma di solidarietà interna a carico degli attuali percettori delle prestazioni. Approfitto di questo punto per aggiungere una nota, non contenuta nella relazione scritta: mi sono permesso di esaminare anche lo stato della situazione per quello che riguarda il servizio sanitario integrativo. Se i contributi sono al di sopra del livello della prestazioni per i senatori in carica, per i senatori cessati dal servizio il livello dei contributi è incredibilmente più basso del livello delle prestazioni. prestazioni. Dato il livello degli assegni vitalizi, qual è la ragione per questa solidarietà al contrario che non capisco? Il livello dei contributi dei cessati dall'incarico dovrebbe essere innalzato in maniera tale da farlo corrispondere al livello delle prestazioni. Non capisco per quale ragione, il livello delle prestazioni e degli assegni vitalizi, si mantenga questa situazione. Non è questa la sede per avanzare specifiche proposte a tale proposito e, soprattutto, io non ho alcun titolo che mi autorizzi a farlo. Era invece mio dovere segnalare la sofferenza finanziaria del sistema (a mio avviso non superata dalle pur rilevanti innovazioni del 1997) e, soprattutto, l'urgenza di un intervento che ci consenta, colleghi, di recuperare credibilità nel rapporto con il Paese.

Questore*. Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente per salutare e ringraziare, anche a nome dei colleghi Comincioli e Thaler in primo luogo il presidente Marini, che, condividendo la richiesta dei senatori Questori, ha voluto che i documenti di bilancio interno fossero sollecitamente portati all'esame del Consiglio di Presidenza prima e dell'Assemblea oggi. Si è così raggiunto, con piena soddisfazione di tutti, quel primo obiettivo, affermato in quest'Aula nel corso del dibattito dello scorso anno, di concludere *l'iter* di approvazione dei documenti di bilancio entro i primissimi mesi dell'esercizio e quindi nel sostanziale rispetto del Regolamento di amministrazione e contabilità, che ne prevede la deliberazione da parte del Consiglio di Presidenza entro la data del 28 febbraio. Saluto ringrazio i Presidenti delle Commissioni permanenti, intervenuti nella riunione dello scorso martedì 27 marzo, e in particolare il presidente Morando per il prezioso contributo recato alla discussione con la sua relazione. Ringrazio, infine, i colleghi presenti e soprattutto quanti oggi interverranno per gli approfondimenti e i suggerimenti che vorranno prospettare. È del tutto evidente che un tale contributo riveste un concreto significato e può ritenersi tale proprio in quanto la partecipazione dei soggetti chiamati a pronunciarsi sui documenti di bilancio, anche attraverso il dibattito odierno in Assemblea, si svolge per la prima volta nelle fasi iniziali dell'anno, rappresentando per i senatori Questori il collegamento più diretto con le esigenze e i problemi della nostra quotidiana attività ed un utile riferimento per gestire il bilancio nell'esclusivo interesse del migliore svolgimento del mandato parlamentare. Il rispetto di termini temporali così ravvicinati sottolinea ulteriormente la portata della rilevante novità regolamentare che ci ha impegnato alla presentazione del rendiconto del 2006 ad appena due-tre mesi dalla sua conclusione. reso possibile da un'intensissima attività delle nostre strutture amministrative. Soprattutto in questo primo anno di applicazione del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità è stato necessario uno sforzo straordinario dei nostri uffici, al cui valore professionale va il nostro apprezzamento. Infatti, insieme ai numerosi e complessi adempimenti contabili e procedurali legati al perfezionamento del consuntivo, si è dovuto negli stessi ridotti spazi temporali predisporre un bilancio di previsione caratterizzato da significative innovazioni. Sono infatti di tutta evidenza le diversità strutturali ma anche stilistiche del progetto di bilancio presentato per il 2007 rispetto ai documenti degli anni passati, talché si è dovuto procedere ad una destrutturazione dello schema espositivo dei bilanci precedenti al fine di rappresentare e mettere a confronto dati comparabili e omogenei. Nel rinviare per gli opportuni approfondimenti alle articolate relazioni che accompagnano i tre documenti di bilancio all'esame dell'Assemblea e riservandomi di esprimermi in sede di replica sugli ordini del giorno presentati, nonché sulle questioni poste dal senatore Morando poc'anzi e da quanti interverranno, mi limito in questa sede a poche essenziali considerazioni. In primo luogo, desidero evidenziare il ruolo che da quest'anno assume il «documento sulle linee guida dell'azione amministrativa» - altra rilevante novità recata dalla riforma del Regolamento di amministrazione e contabilità in relazione alla gestione del bilancio interno. Recependo le indicazioni emerse dal dibattito in proposito svoltosi nella riunione del Consiglio di Presidenza dello scorso dicembre, l'indice del prodotto interno nominale recato dal Documento di programmazione economico-finanziaria per cento è stato assunto come limite alla crescita delle risorse complessive iscritte a bilancio e quale parametro di riferimento per la missione di contenimento della spesa per l'intero triennio 2007-2009 e anzi siamo rimasti leggermente sotto tale limite, attestandoci al 2,7 per cento. Come si è già detto nella relazione di accompagnamento, tale missione - in aggiunta al taglio di 23 milioni di euro sul bilancio 2007 rispetto alla dotazione originariamente richiesta - è testimone eloquente dell'attenzione posta dal Senato all'esigenza di risanamento della finanza pubblica. Desidero inoltre sottolineare come i senatori Questori, confermando la linea di rigore e di trasparenza che tradizionalmente caratterizza i nostri bilanci interni, hanno voluto che gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa rappresentassero in maniera diretta le decisioni programmatiche e i conseguenti piani di esecuzione assunti dalla Presidenza e dal Collegio dei senatori Questori. In questa specifica direzione, di immediata e piena conoscibilità della spesa già pianificata, vanno lette le tabelle analitiche contenenti gli impegni contrattuali già operanti sulla spesa del 2007, che si possono consultare in allegato al progetto di bilancio secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità. Lo scorso anno, come risulta dal rendiconto di esercizio, nel settore delle spese di natura corrente non obbligatoria abbiamo realizzato risparmi di oltre 5,7 milioni di euro. Il dato, anche se in parte riconducibile alle minori esigenze che normalmente si registrano in un anno di cambio legislatura rispetto ad un anno di piena attività, è significativo di una politica virtuosa costantemente perseguita dai senatori Questori e dalla Presidenza nella gestione del nostro bilancio. Anche quest'anno, e concludo, intendiamo raggiungere qualche positivo risultato in termini di economia e di risparmio, senza comunque incidere sulla qualità e l'ampiezza dei servizi necessari al pieno svolgimento del nostro mandato, la cui piena efficienza rimane l'obiettivo prioritario della nostra azione amministrativa. Così pure ci sentiamo impegnati in prima persona a garantire la necessaria copertura finanziaria di specifici obiettivi programmatici esposti nel documento sulle linee guida dell'azione amministrativa, ed in particolare alla definitiva soluzione del problema degli spazi, sul quale in sede di replica fornirò ulteriori elementi di valutazione e di conoscenza. onorevoli colleghi, non posso non iniziare queste brevi riflessioni se non manifestando apprezzamento al presidente Marini proprio per quanto ha detto poco fa il collega Questore Nieddu, nel senso che registro anch'io con soddisfazione il fatto che quest'anno, dopo molti anni, dibattiamo il bilancio preventivo del Senato nei tempi appropriati. Ricordo che nel passato

Per quanto abbiamo ascoltato poco fa, dico subito che sottoscrivo la relazione del senatore Morando, che ha toccato problematiche in gran parte condivisibili. Vorrei dare il mio contributo

Senato (presidente del Senato era allora il senatore Nicola Mancino), ridisegnando la mappa della funzioni e degli uffici del Senato raggruppandoli in tre grandi aree di coordinamento ed ammodernando così la struttura, proprio come nel Paese si chiedeva. Si discuteva molto della necessità di modernizzare il sistema burocratico del nostro Paese, e si fece proprio nella legislatura dal 1996 al 2001, convinti e consci che l'ultima riforma organica del Senato venne fatta da un grande uomo politico, l'indimenticabile presidente Amintore Fanfani, che venti anni prima, per la prima volta dopo il 1948, aveva messo mano all'organizzazione del Senato proponendo e suggerendo modifiche veramente organiche e funzionali. Nella legislatura che va dal 1996 al 2001 si mise mano alla cosiddetta riforma Fanfani, procedendo con istituti nuovi. Lo voglio dire perché - lo sanno bene i colleghi della struttura che io per primo stimo, e ricordo con favore l'esperienza di quella legislatura - per la prima volta furono, ad esempio, organizzate gare con inserzioni sui giornali; il Senato si aprì all'esterno. Per non dire, poi, della selezione per merito per arrivare alla carica di dirigente. Nel Senato, prima di allora,

Un aspetto è quello della riforma previdenziale del personale. Noi abbiamo - è bene dirlo e ribadirlo in questa sede - un personale di alta qualità. Al Senato è difficile accedere, ma il livello dei nostri dipendenti - dirigenti, funzionari e quant'altro - è di elevata qualità,

di grande qualità, dove lavorano persone capaci, professionalmente attrezzate, adeguatamente motivate, esistono 13-14 sigle sindacali. Questo non l'ho mai capito. Ripeto, l'esistenza di 13 sigle sindacali nell'istituzione chiamata Senato non l'ho mai capita. Credo che questo sia il motivo - lo dico *a posteriori*

So che è difficile fare la controparte del sindacato, però l'esperienza credo sia utile per dire che ormai i tempi sono maturi per superare questa anomalia.

della nostra istituzione alla realtà esterna attraverso un processo graduale che rispetti i diritti acquisiti ma che, al contempo, introduca le logiche che si vogliono inserire a livello di sistema previdenziale complessivamente considerato. La seconda questione mi interessa ancora di più. È una riflessione che voglio fare in termini politici, assumendomene la responsabilità, ma con una ricaduta sulle questioni interne. nel Paese una tendenza a privilegiare la governabilità - mi rivolgo al collega Manzella che di queste tesi è sempre stato

In un contesto che vede le situazioni a cui prima facevo riferimento, è ovvio che le istituzioni chiamate ad esercitare un ruolo e una capacità di produrre un indirizzo politico debbano essere strutturalmente organizzate perché i singoli parlamentari e i Gruppi parlamentari

(facciamo le indagini e non solo non abbiamo i pochi euro per permetterci consulenze esterne ma non abbiamo una struttura tale da contrastare ciò che ci viene dall'esterno e quindi siamo sempre più deboli di fronte all'offensiva di *lobby* variamente organizzate);

Signor Presidente,dobbiamo realizzare questa convergenza e mi sembra che in tal senso lo stesso senatore Morando ha ricordato che nell'ultima finanziaria, nell'ultima finanziaria, nell'enorme quantità di commi, ce ne sono un paio che meritano l'attenzione del nostro Collegio dei Questori, laddove si afferma che per

non sono coriandoli, ma risorse piuttosto robuste che, a parer mio, vanno finalizzate per dotarsi in modo serio di questa strumentazione che mi sembra molto importante. Pertanto sono assolutamente d'accordo, anzi immagino che si possa fin d'ora ipotizzare una fusione degli apparati serventi, perché le gelosie

che esistono degli interessi comuni che vanno individuati e messi a regime, immaginando che, ancora di più di quanto è stato fatto quest'oggi, possano procedere nella collegialità di una direzione che significa: facciamo assieme un certo lavoro e produciamo lo stesso lo stesso risultato. Sulla questione del personale insisto perché perché è veramente un equivoco. Do atto che il Collegio dei senatori Questori ha fatto finora il possibile per contenere le spese e procedere nella logica di una politica di rigore,

Credo che i colleghi dovrebbero conoscere bene la riforma del 1997, che fu una riforma seria.

è falso. Con la riforma del 1997 nessun parlamentare, compreso il sottoscritto che ha partecipato a sei legislature, può andare in pensione prima di aver

la riforma del 1997. Lo dico al Collegio dei Questori perché mi sento personalmente e moralmente un po' ferito. Per cortesia, applicate integralmente la riforma del 1997, perché mi risulta che soprattutto per il protagonismo della Camera alcuni istituti che andavano nella direzione di introdurre norme severe e serie sono stati messi sul binario morto, nel dimenticatoio. Andate a leggere le disposizioni approvate dal Collegio dei senatori

identica a quella del nostro Paese. Qual è il motivo per cui in Italia, diversamente dai francesi e dagli inglesi, anziché discutere di problemi sostanziali si discute della riduzione del numero dei parlamentari? Non vorrei che si facesse lo stesso sulle pensioni vitalizie dei senatori. Discutiamone, introduciamo norme ancora più rigorose, ma

che vede una netta distinzione, anzi una assenza di regolamentazione, per tutto il personale assunto a partire dal 1998. Comunico all'Aula e ai relatori che il Consiglio di Presidenza è stato convocato per il giorno 17 aprile

*(Aut)*. Signor Presidente, signori Questori, intendo innanzitutto esprimere un vero apprezzamento per i servizi forniti dal Senato, dalla Presidenza e specialmente dai nuovi impulsi provenienti dal Collegio dei senatori Questori, che non sono solo soddisfacenti, ma ottimali. Il mio giudizio positivo vuole soffermarsi in particolare sui servizi con i quali noi senatori abbiamo un contatto diretto, senza con questo voler diminuire il valido contributo di tutti gli altri servizi forniti, che però forse conosciamo un po' meno. La Presidenza, l'Aula,

Nell'ambito degli obiettivi per il 2007, condividiamo pienamente la scelta della Presidenza e dei senatori Questori di contenere il più possibile le spese. Mi congratulo con quanto è stato poco fa annunciato dal senatore Nieddu

così come trovo opportuna la decisione di potenziare l'informatizzazione con tutta una serie di supporti per i senatori e i dipendenti che, di fatto, hanno come obiettivo il risparmio dell'uso della carta.

Infine, sono d'accordo anche con l'intento di porre in essere il *turn over* del personale, nonché la riorganizzazione degli uffici. Signor Presidente, mi consenta di fare ora una riflessione in materia di informazione e *mass media*.

la nozione del vero lavoro del Parlamento e degli apporti di proposte provenienti dai loro rappresentanti. Non si tratta di un problema di visibilità. Lo sottolineo perché noi tutti abbiamo nel nostro collegio la possibilità di attivarci e ricevere la necessaria attenzione dai *media* locali. piuttosto, della valorizzazione di uno dei tre poteri della democrazia: quello legislativo, accanto al potere giudiziario e a quello esecutivo.

che nella scorsa legislatura, in sede di discussione del bilancio interno del Senato, avevo presentato un ordine del giorno firmato trasversalmente da oltre un centinaio di colleghi, in cui si faceva presente questo *deficit*, non solo e non tanto di informazione, quanto piuttosto di democrazia e pluralismo dell'informazione, chiedendo alla Presidenza e ai senatori Questori che si attivassero per supportare maggiormente un servizio che mettesse

oltre cento senatori di maggioranza e opposizione, che concordavano sull'obiettivo. In esso si dice che i *mass media* spesso trascurano i lavori dei singoli parlamentari, i loro interventi e le loro proposte, sia in Aula e soprattutto nelle Commissioni, il lavoro di sindacato ispettivo, che invece dovrebbero essere valorizzati mettendo in evidenza anche il lavoro di chi non ricopre posizioni di rilievo a livello nazionale. Ciò, per esempio, viene fatto da anni da qualche agenzia parlamentare in grado anche di produrre servizi audiovisivi divulgativi del lavoro dei parlamentari.

indicati. Un'agenzia che ha svolto e tuttora svolge questo capillare servizio era, tra le altre, tutte preziose, l'AgenParl,

sulla scorta della nostra richiesta presentata in Aula. Il contratto però è scaduto e purtroppo non è stato più rinnovato.

La questione di fondo - ribadisco - non è quella di una nostra particolare visibilità nella società della comunicazione, bensì di far conoscere alla maggioranza dei cittadini il cuore dell'impegno più serio del nostro lavoro, che

con il proprio elettorato, le pratiche relative al proprio collegio. Il lavoro è molto intenso, ma l'opinione pubblica pensa esattamente il contrario. Mi auguro Mi auguro pertanto che il Collegio dei senatori Questori e il Consiglio di Presidenza tengano conto di questa riflessione e, compatibilmente con le risorse a disposizione e la necessità di ridurre le spese, che avevo sottolineato e che condivido pienamente, garantiscano il pluralismo nell'informazione e lo favoriscano la pluralità dei mezzi di informazione presenti in Senato. Ringrazio il Presidente, i senatori Questori e tutto il personale coinvolto in questo lavoro di supporto.

della democrazia parlamentare nel nostro Paese. Esprimendo adesione completa alle

l'apporto della biblioteca. Quindi, è un augurio che si sia cominciato dalla fusione delle biblioteche. Questa idea di un'area consorziale è ancora più pregnante nella prospettiva di una modificazione strutturale del nostro Senato: quando si sarà sviluppata quell'idea di «base regionale» che è già nella nostra Costituzione e quando si sarà realizzato un bicameralismo differenziato, bicameralismo differenziato, allora tanto più sarà necessario che le Camere abbiano questo filo comune documentario che le unisca - mi si scusi l'espressione - in una dimensione nazionale, nel senso parola. Andiamo ora all'ordine del giorno, che è stato firmato dai 14 Presidenti di Commissione. Credo che sia un fatto inedito nella piccola storia di questa

si ritorni alla centralità del lavoro di Commissione in questa Assemblea: centralità del lavoro di Commissione che, come si sa, segna il punto preciso del passaggio dalla premodernità

nel suo libro «Stato e rivoluzione», quando capisce che c'è una evoluzione dei parlamenti in un'articolazione in commissioni specializzate dice: «Attenzione, i parlamenti borghesi si stanno trasformando da mulini di chiacchiere in luoghi di lavoro». Vede,

delle corporazioni, si capì che, anche in quel momento, occorreva creare un luogo di lavoro. Le Commissioni della Camera dei fasci e delle corporazioni, come attesta Renzo De Felice, dettero del filo da torcere al Governo di allora. I disegni di legge del

direi precipuamente, sulla valorizzazione del lavoro di Commissione. Allora si disse, infatti, che le Commissioni non avevano solo il compito referente dell'articolo 72 della Costituzione, ma dovevano avere anche un compito di controllo, attraverso le interrogazioni

conoscitivo, aprendo il Parlamento, che fino a quel momento era coartato nel rapporto bilaterale Governo-Parlamento, a quelle che si dicono le espressioni della società civile: nascono le indagini conoscitive. Ecco quindi che, per opera di Sandro Pertini

perno del nostro vivere civile così come lo concepisce la modernità. Ma la vera norma della democrazia parlamentare è il cambiamento, è l'adesione a quelle che sono le necessità

cittadini. Ecco perché 14 Presidenti di Commissione hanno firmato questo ordine del giorno. Perché la situazione non è più tollerabile in quanto ne va non solo della funzionalità tecnica della nostra Assemblea, ma della stessa democrazia parlamentare, ripeto, che vuole il confronto vero e non fittizio né tribunizio. Perché poi di questo si tratta: di un parlamentarismo tribunizio, quando ci confrontiamo gli uni contro gli altri in una tribuna meramente meramente propagandistica, sapendo che poi il senso delle nostre decisioni è precondizionato e comunque non modificabile. Costringiamo così la partecipazione cittadina, perché certo queste riunioni interstiziali non possono avere

al recente dibattito svolto in quest'Aula sulle questioni ambientali e i cambiamenti climatici. Voglio richiamare quel dibattito, perché

produttivi indicando obiettivi da raggiungere (in generale, sapete perfettamente che la Commissione europea ci ha dato l'indicazione

anche se - questo farà parte del mio intervento in dichiarazione di voto - è evidente che in generale tutto il capitolo delle spese non obbligatorie ha avuto un contenimento ed il bilancio 2007 opera comunque nel rispetto del 7,7 per cento. Però, è assolutamente fondamentale da parte nostra, dell'Amministrazione del Senato e dell'Assemblea far sì che tra i diversi interventi, volti a contrastare il cambiamento climatico, quindi per il risparmio energetico, vi sia anche una assunzione di responsabilità da parte del Senato:

È necessario per questo - tale è il senso dell'ordine del giorno - presentare un progetto di efficientamento energetico, efficientamento energetico, che contiene in sé sia tutte quante le azioni di programmazione, di pianificazione, di progettazione e di realizzazione che consentono appunto di raggiungere l'obiettivo del risparmio di energia. Già nel corso

È necessario anche - sapete che anche molte imprese private - un po' meno purtroppo nell'amministrazione pubblica, ma su questo ci si sta impegnando - stanno indicando delle figure

un progetto di efficienza energetica che ci faccia conseguire già entro il 2007 delle riduzioni significative, ma anche di individuare una figura all'interno della struttura, che può assumere su di sé la responsabilità dell'efficienza energetica dei palazzi e delle strutture del Senato, quindi attraverso la nomina e l'individuazione di un *energy manager*. Il secondo ordine del giorno ha a cuore le stesse problematiche. Vorrei anche ricordare che che all'interno della finanziaria al comma 1108, dell'articolo 1, non solo si sono date delle indicazioni ma addirittura vi è anche un altro comma che dà delle indicazioni a tutto il capitolo degli acquisti della pubblica amministrazione, indicando il parametro della sostenibilità anche per gli acquisti.

la sostenibilità ovviamente non solo sulle questioni energetiche, ma più complessivamente anche le norme di sostenibilità sugli acquisti della pubblica amministrazione sono assolutamente fondamentali perché anche questi ci aiutano a conseguire l'obiettivo che ci siamo prefissi di una riduzione in tempi rapidi delle emissioni. Tra l'altro, ormai è sempre più diffusa l'applicazione nelle pubbliche amministrazioni dei *green public procurement*, che significa appunto la possibilità

enorme - una leva fondamentale per determinare anche un'adeguata sensibilità del mercato alla sostenibilità ambientale. ambientale. Vorrei ricordare, fra l'altro, che il settore degli approvvigionamenti pubblici rappresenta mediamente il 12 per cento del prodotto interno lordo dell'Unione Europea e raggiunge il 17

si possano riorientare gli acquisti e il Senato possa quindi trasferire la propria capacità di acquisto su prodotti a impatto ambientale ridotto, includendo criteri ambientali nelle procedure di acquisto. Ciò significa che anche che anche nei capitolati delle gare di appalto debbono essere indicati innanzi tutto i criteri ambientali e che il Senato deve avere concretamente la possibilità di ridurre gli impatti delle proprie attività, incrementando la domanda per i prodotti sostenibili sostenibili e contribuendo a sospingere le imprese a produrre beni con migliori prestazioni ambientali. Se ne

Quindi, chiediamo che il Collegio dei senatori Questori nel predisporre le gare introduca adeguati livelli di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto per beni e servizi, anche al fine di favorire la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di limitare, sostituire ed eliminare l'acquisto di prodotti con un impatto elevato dal punto di vista ambientale. Vi è poi la questione della raccolta differenziata. Questo è il luogo principe di un uso, di un consumo e anche di un abuso

il 31 dicembre 2011. Credo che il Senato per primo debba contribuire al raggiungimento di tali percentuali. Chiediamo e quindi ovviamente al Consiglio di Presidenza, di introdurre rapidamente tutte le adeguate procedure atte ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti, in primo luogo della carta, perché, torno a ripetere, è veramente incredibile

Signor Presidente, tenterò di dare l'esempio svolgendo un intervento sicuramente al di sotto dei venti minuti che mi hanno assegnato, anche perché, non essendo un tecnico di questo tipo di materie, debbo solo rallegrarmi innanzi tutto con il relatore, il presidente Morando, per l'illustrazione che ha fatto a tutti noi della situazione, e il controcanto, diciamo così, che ha fatto, il che potrebbe risolvere l'intero dibattito per quanto riguarda la sua parte contenutistica. Desidero anche ringraziare in questa circostanza i colleghi Questori, che con impegno personale sicuramente degno di lode ci aiutano a lavorare meglio, rappresentano le nostre esigenze presso il Consiglio di Presidenza, e anche il Consiglio di Presidenza. Non perché nei periodi di Natale e Pasqua si diventi più buoni, ma con sincero spirito di gratitudine desidero ringraziare la Presidenza e tutto il personale per l'impegno che profondono nell'esercizio della loro professione, della loro carica istituzionale, che consentono credo al Senato di dare una buona immagine di sé soprattutto all'interno. Questa precisazione motiva la vera ragione per la quale ho chiesto di intervenire: tutto ciò si risolve generalmente in un discorso tra noi. Se debbo segnalare una carenza relativamente ai lavori del Senato è la scarsa capacità di pubblicizzazione di quanto avviene in quest'Aula verso l'esterno, vale a dire verso i cittadini che in questo momento, diciamocelo francamente, non hanno una concezione al massimo dell'entusiasmo per quanto riguarda il lavoro delle istituzioni politiche e parlamentari. Sarebbe opportuno, allora, prevedere qualche forma di informazione, di sensibilizzazione, di coinvolgimento più concreta per aiutare il cittadino a conoscere per poter poi giudicare con maggiori argomenti in mano. A tale proposito mi piace fare un confronto con quanto accade in un'istituzione che sotto questo aspetto è sicuramente esemplare e all'avanguardia: il Parlamento europeo.

silenziosa, ma attenta, di visitatori. Qui oggi non vedo una persona in tribuna, eppure era una giornata favorevole con le vacanze di Pasqua. Al Parlamento europeo c'è un sistema di visite che costantemente, in maniera ordinata, attenta, ma aperta a tutti, vorrei dire democratica, per usare un termine perfino banale, consente al cittadino di toccare con mano l'istituzione, quanto sta accadendo, e soprattutto di essere testimone fisico di come si lavori e di quali temi vengano trattati. Mi pare che il nostro Senato non abbia questa attenzione con la dovuta convinzione: lo dico anche perché in un anno da che sono qui ho chiesto cinque volte di poter far entrare dei gruppi di visitatori e per cinque volte mi è stato detto che non era possibile,

di poter far conoscere il luogo in cui lavora o si esprime ai propri elettori non riesca ad avere la possibilità di far passare un gruppo. E allora mi chiedo come facciano al Parlamento europeo (che vede la presenza di oltre 700 parlamentari e 27 Paesi) dove, costantemente, durante le plenarie di Strasburgo, nella settimana di lavoro, ma anche durante le tre settimane di lavoro a Bruxelles, è garantito l'ingresso di centinaia di gruppi di visitatori, ordinati e condotti da

i funzionari illustrano ai cittadini le modalità attraverso le quali i parlamentari esercitano il loro mandato. Spiegano il mandato democratico. La mia richiesta, amorevole ma ferma, è pertanto quella di rivedere le norme che ispirano questo tipo di apertura che esiste - lo so - anche qui in Senato, ma forse con procedure un po' troppo restrittive, limitative.

entrare al Senato. Quinto assalto e quinta sconfitta. Perdonatemi, ma un pochino di animosità me la sento addosso perché mi vergogno un po'. Non conto proprio niente, debbo dire ai miei elettori. Non riesco nemmeno a farli entrare. Per passare dalla protesta banale, alle proposte costruttive, aboliamo un po' di burocrazia, apriamo di più queste porte, consentiamo turni più fitti. Il personale è molto bravo; io l'ho ascoltato mentre ad alcune scolaresche spiega ed illustra le bellezze di questo palazzo. Ma non basta nemmeno questo. Così come accade al Parlamento europeo - se c'è un modello buono, non vergogniamoci a copiarlo - bisogna che questi visitatori siano messi anche in condizione di incontrare il proprio senatore, di ascoltare in una relazione serena l'attività che viene svolta. Occorre quindi prevedere una sala nella quale sistemare i visitatori e avere quella mezz'oretta di contatto che dà anche un senso alla visita. Non oso intervenire sul piano finanziario, anche se non sarebbe male, sempre prendendo l'esempio di Bruxelles e Strasburgo, consegnare nelle mani di questi visitatori un *gadget* qualsiasi, di valore simbolico, che ricordi il passaggio nelle sale del Senato. Il costo non dovrebbe essere straordinario. Dopo aver ascoltato la relazione sul bilancio non oso, presidente Morando, immaginare di proporre quello che già esiste al Parlamento europeo, dove ogni parlamentare ha due viaggi all'anno finanziati dal Parlamento. Ogni anno due gruppi di visitatori sono finanziati, per ogni deputato, dal Parlamento stesso. sono poi altre forme attraverso le quali il parlamentare può contribuire al finanziamento dei gruppi, perché là si crede veramente al valore di questo incontro ravvicinato che esprime non solo un gesto di simpatia, ma un'occasione di trasparenza che non dobbiamo mai dimenticare. Quindi, sotto il profilo delle aperture democratiche e della pubblicizzazione, questa mi sembra una proposta che si possa prendere in esame. So qual è la risposta che mi date perché già è stata data in privato: qui le regole sono così; qui non si fa come al Parlamento europeo, non si è mai fatto. Tuttavia, il coraggio di una riforma, Presidente, bisogna averlo ad un certo punto. Se c'è un modello valido che in dimensioni macroscopiche, come quelle del Parlamento europeo, funziona e dimostra di essere molto gradito al cittadino, perché non provare con le nostre forze ad imitarne gli effetti positivi? Avrei voluto concludere qui il mio intervento, ma l'intervento del presidente Marini mi ha rassicurato su un tema che comunque avevo intenzione di toccare con tutta la prudenza del caso, ovvero quello della condizione normativa, salariale e previdenziale del personale del Senato. Dopo appena un mese di lavoro qui dentro fui avvicinato anch'io, come credo molti altri colleghi, da alcuni dipendenti che mi dimostrarono una situazione imbarazzante per un'istituzione come il Senato, dove più o meno il 50 per cento dei dipendenti ha una forma di rapporto ispirata al precariato più che alla sicurezza. Il Presidente poco fa ha detto che è intenzionato ad intervenire, che ha già le misure da proporre e quindi mi metto in attesa e in ascolto delle soluzioni che saranno trovate

di personale in attività qui al Senato. Ho una cartella con una serie di nomi, cognomi e situazioni che ho già consegnato tra l'altro ai Questori. Quindi, prima di parlare degli assistenti parlamentari, che rappresentano da sempre un caso molto delicato, vediamo di sistemare queste persone.

dall'intervento del collega Grillo, che ha toccato un tema molto delicato che in questi giorni è rimbalzato ancora una volta su tutta le stampa nazionale, in modo particolare, con una violenza inaudita, sulla stampa della mia Regione, il Trentino-Alto Adige

credo che dobbiamo cercare di fare trasparenza anche sotto questo aspetto. Forse per contribuire a far capire che abbiamo una certa disponibilità a ragionare, attirandomi sicuramente l'antipatia *bipartisan* di tutta quest'Assemblea, e probabilmente anche di chi sta fuori, sono d'accordo sul fatto che il trattamento pensionistico dopo una legislatura legislatura sia difficilmente proponibile a chi ha un lavoro normale e deve attendere 30-35 anni per maturare la pensione. Credo però che sia anche un istituto superato dai tempi, faccio una proposta concreta per dimostrare che non vengo qui a fare della vuota demagogia: quando un cittadino viene eletto ad una carica parlamentare non ha bisogno di un trattamento pensionistico ulteriore, perché si immagina che faccia parte già di una categoria professionale che preveda per lui pensione, stipendio, previdenza e assistenza come tutti. Allora, perché non istituire una sorta una sorta di staffetta per cui ogni cittadino che diventa parlamentare conserva e si porta dietro il proprio trattamento previdenziale, non solo, ma anche il proprio livello stipendiale

professionale e personale. In questo modo, tra l'altro, terminato il mandato non vi sarebbero scossoni al rientro nel proprio lavoro. So che la proposta è impopolare, soprattutto per chi vede nel mandato parlamentare un miglioramento della propria situazione, ma se vogliamo essere trasparenti e coerenti è una proposta realistica. aggiungere un momento d'imbarazzo che provo quando i cittadini mi chiedono se il nostro lavoro qui sia obbligatorio o facoltativo. Molti nostri colleghi, infatti, non esitano a dimostrare anche pubblicamente di continuare a svolgere anche la loro attività professionale, soprattutto certe professioni che vengono alla luce del sole. Io ero dipendente pubblico - giornalista RAI - e non ho avuto neanche il tempo di scegliere: il giorno dopo l'elezione, nel 1994, fui messo in aspettativa.

certo, come ho detto in apertura, di attirarmi in questo modo l'antipatia e l'opposizione di tutti, ma credo che quando i cittadini ci eleggono parlamentari ci chiedono anche di avere il coraggio di attingere da un serbatoio che è molto lontano da quello che quotidianamente alimenta il nostro modo di proporci, cioè da quello della verità e delle convinzioni più intime. Avevo dentro questi ragionamenti da molto tempo e - guardate un po' - un semplice bilancio del Senato mi consente di portarli alla vostra considerazione e io credo di poterli proporre alla riflessione dei benpensanti, naturalmente assieme a tanti auguri di buona Pasqua. *(UDC)*. Signor Presidente, signori Questori, senatori, è stato mantenuto l'impegno di assicurare il dibattito in Assemblea e la relativa deliberazione nei termini adeguati e tali da rispettare il suo ruolo previsivo. necessario riflettere innanzitutto sul ruolo dell'istituzione Senato e sulla sua funzionalità. Non vi è dubbio che esso riflette le difficoltà derivanti dal risultato elettorale con una sostanziale parità e dal ruolo determinante assunto dai senatori a vita. Tutto ciò sta determinando la surrettizia affermazione di un monocameralismo che potremmo definire imperfetto. A tale riguardo ho presentato una proposta di modifica del Regolamento del Senato per evitare che i senatori a vita siano trascinati nell'agone politico e mantengano quel ruolo così come individuato dai Costituenti. È pur vero, signor Presidente, che tra gli stessi Costituenti l'idea dell'onorevole Alberti come presentatore era di assicurare ai sommi, ai geni tutelari della Patria, una tribuna che essi non avevano. Egli affermò incautamente che i senatori a vita, proprio per il loro esiguo numero, «non potranno mai in nessun modo spostare il centro di gravità di una situazione politica in Senato». Mai affermazione fu - per così dire - contraddetta. Costituzione nasce, dunque, su iniziativa dell'onorevole Alberti, il quale osservò che per quanto attiene al primo comma «si tratta di ricollocare nel Senato personaggi i quali non solo hanno simboleggiato, ma hanno sintetizzato dei periodi politici, perché il Presidente della Repubblica è il tipico rappresentante riassuntivo di questa sintesi». Tale proposta fu accettata - sappiamo com'è andata - considerando che i Presidenti della Repubblica, per il posto che hanno occupato, «non possono riscendere dal loro mandato nell'agone Così non è, perché i senatori di diritto e a vita, a differenza del passato, stanno giocando e giocano un ruolo squisitamente politico, diventando arbitri della sorte di una maggioranza. La questione non è secondaria e dovrebbe essere affrontata in termini costruttivi e senza posizioni preconcette. Mi rivolgo in particolare ai senatori Manzella e Maccanico, così attenti a tali vicende. Nei fatti, poi, la posizione dei senatori di diritto e a vita è oggi strettamente legata a quella del Gruppo Misto, al quale aderiscono, con la conseguenza di sottostare alle direttive politiche della Presidenza di tale Gruppo. La posizione dei senatori a vita, senatore Manzella, si scontra con la collocazione nel Gruppo Misto, ponendo seri problemi sia all'attività del Gruppo, sia rispetto alla posizione individuale degli stessi senatori a vita. La fonte della loro legittimazione è sostanzialmente diversa da quella dei senatori eletti. Va poi segnalata l'anomalia dei senatori a vita che nei lavori di Commissione vengono sostituiti meccanicamente da componenti del Gruppo Misto, venendo meno all'espressione più autentica della loro posizione, che risiede proprio nel fatto di avere illuminato la Patria per altissimi meriti. Non si può delegare la loro presenza nei lavori quotidiani di Commissione. Credo che sarebbe opportuna una modifica dell'articolo 14 del Regolamento, nel senso di rafforzare e salvaguardare la loro posizione in modo più autonomo rispetto alle funzioni di indirizzo politico del Senato,

(siamo più rivolti a problemi esterni che non a quelli veri dell'istituzione Senato). Tutto ormai viene affrontato in prima lettura alla Camera e al Senato viene assegnato un ruolo residuale, diventando spesso solo luogo di ratifica. Lo abbiamo visto anche ieri: mi sono rifiutato

Non viene neppure esaltato lo strumento del sindacato ispettivo, in particolare il *question time* su questioni di grande attualità, che potrebbe determinare una forte visibilità e centralità del Senato.

La sessione di bilancio, Presidente, ha dimostrato l'assoluta incapacità per il Senato di disporre dei dati di bilancio. Nonostante ogni buona volontà, ad oggi non abbiamo i resoconti stenografici della sessione. Il presidente Morando si era impegnato: sicuramente non sarà come in passato, avrete i resoconti stenografici. Questo si rifletteva anche sulla stesura dei resoconti, i quali venivano fatti come verbale di Commissione, senza alcun approfondimento. Tutto questo è mancato.

Il collegamento con la Ragioneria generale dello Stato, che fu un grandissimo risultato raggiunto per la caparbietà dell'onorevole La Loggia *senior*, allora presidente della Commissione bilancio della Camera, richiede un'ulteriore fase di ristrutturazione, dotando il Parlamento di mezzi e strumenti in grado di riequilibrare quel rapporto Governo-Parlamento che si è progressivamente alterato. Queste cose non le sostengo solo oggi, Presidente, ma anche quando il ministro dell'economia era Tremonti. L'intercameralità di alcuni Servizi come la biblioteca e l'archivio storico è cosa certo più facile e in grado di produrre risparmi di spesa.

Più difficile è l'unificazione del Servizio bilancio, senza minare l'autonomia di ciascuna Camera, senza modificare le norme costituzionali sul bicameralismo. Non vorrei che si guardasse più alla forma che alla sostanza. Di qui la necessità di determinare le condizioni, senatore Manzella, per l'*on line* sulle entrate e sulle uscite fiscali. È davvero curioso che, mentre per il cittadino, per il commercialista, per l'esercente arti e professioni, per ogni esercizio commerciale si afferma l'*on line* sia nelle dichiarazioni dei redditi che nei flussi di gestione quotidiana il Parlamento resti fuori da questo processo di avanzamento. A tale riguardo, signor Presidente, non ho condiviso né la scelta fatta nella manovra finanziaria di avere una dotazione di 600.000 euro per il Servizio bilancio, né quella sostenuta dal Presidente della Commissione bilancio e relatore di questo provvedimento - ancora assente di un concorso specialistico per integrare le risorse umane di questo Servizio. Trovo davvero singolare che, rispetto ad un avanzo di gestione di 42 milioni di euro (tra l'altro spalmato in due esercizi, contro il Regolamento di amministrazione e contabilità, il cosiddetto RAC, e senza alcuna ragione plausibile, sia perché l'intera somma poteva essere traslata sull'intero esercizio successivo, in adesione appunto al RAC, sia perché per eventuali evenienze, rispetto ad eventuali ritardi, si poteva fare affidamento sul conto di riserva), sia arrivati alla decisione di questa dotazione supplementare veramente risibile. Tutto poteva essere fatto all'interno delle poste di bilancio senza minarne l'autonomia, mentre andiamo a toccare il principio di autonomia dei fondi del Senato. Se vogliamo veramente rafforzare la capacità di verifica e di valutazione dei dati di bilancio è necessario acquisire professionalità mature, come quelle presenti in enti, centri di ricerca, strutture specialistiche dello Stato, in grado di fornire adeguate valutazioni critiche che un neolaureato non può determinare. Abbiamo bisogno di professionalità di alto profilo, inquadrate all'interno di un Servizio, quello del bilancio, senza creare strutture alternative e parallele. Lavia migliore, a mio parere, è quella delle consulenze di altissimo profilo, così come sarà fatto per il 2007, che assicurino un risultato elevato e, al tempo stesso, garantiscano la dovuta flessibilità, senza quelle rigidità che invece si vogliono rimuovere soltanto a parole. Non si comprende allora perché la soluzione transitoria ipotizzata per il 2007 non debba essere perseguita anche per il futuro. Ritengo di sottoporre ancora una volta la possibilità di introdurre il controllo di gestione, per il quale mi sono inutilmente speso, da solo... *(Commenti del Chiedo scusa, c'era anche il senatore Viespoli che mi ha affiancato in questa richiesta. Questo rappresenta lo strumento più adeguato per una sana ed efficace gestione amministrativa. Non posso non evidenziare due questioni. La prima riguarda la mancata soluzione della rilevante problematica previdenziale, che assume ancora un più forte significato rispetto al numero di concorsi programmati, che vanno ad appesantire l'irrisolta questione per i dipendenti entrati in ruolo dopo il 1° gennaio 1998, creando un'insofferenza nel personale che è diventata ormai si tocca con mano, in presenza di un passaggio al regime contributivo per un numero rilevante di persone. La questione va affrontata e chiusa rapidamente, com'è negli auspici espressi poc'anzi dal Presidente e da tutti noi. Va attentamente valutata la dinamica di crescita del personale, che ha raggiunto nell'ultimo quinquennio una percentuale del 30,84 per cento, passando da 830 a 1.086

l'altra questione sulla quale mi sarei aspettato una qualche attenzione da parte del presidente Morando concerne il contributo indiretto da parte del bilancio dello Stato al fondo CAI. È un fondo assicurativo individuale, peraltro

La tabella allegata al bilancio interno dimostra che c'è un rilevante intervento sul conto economico e che i contributi dunque non coprono l'intero volume delle spese. Per quanto riguarda la politica di investimento, occorre salvaguardare la spesa per l'informatica, riconsiderare alcune scelte relative alla politica degli spazi, anche perché particolarmente costose, e un urgente piano di azione rispetto alla modernizzazione degli ascensori (mi sono permesso di

e non i ritardi fin qui registrati. Mi preme anche sottolineare che è assai discutibile la scelta di distribuire l'avanzo dell'esercizio 2006 tra gli anni 2007 e 2008 perché in tal modo, onorevoli Questori, si contraddice lo schema previsto dal nuovo regolamento di contabilità: approvazione del rendiconto dell'anno precedente e del preventivo dell'anno corrente. Trasferendo una parte cospicua al secondo anno successivo a quello in cui si è realizzato l'avanzo, infatti, non si ha modo di apprezzare la continuità tra gli esercizi di bilancio, come avviene, invece, nei bilanci societari. In un sistema contabile aziendale, infatti, il fondo di cassa finale (che nel caso del Senato corrisponde all'avanzo di esercizio) rappresenta anche il fondo iniziale dell'esercizio successivo. Operando nel modo proposto, inoltre, si produce l'accantonamento di una somma «fuori bilancio» di oltre 26 milioni di euro, pari a circa il 4,5 per cento del complesso delle entrate. Questo importo, viceversa, avrebbe dovuto correttamente essere impiegato per ridurre di pari importo la dotazione ordinaria, proprio in quello spirito di contenimento della spesa pubblica di cui si parla più volte nei documenti. In merito ai rendiconti si osserva che le relazioni di accompagnamento, mentre si diffondono sull'attività amministrativa e di documentazione, poco o nulla dicono sulla composizione delle entrate, in particolare su quelle diverse dai trasferimenti dello Stato, come i redditi patrimoniali, e se essi derivino solo da interessi sui conti correnti o da altro tipo di investimenti, ovvero sulle partite di giro e i movimenti di cassa (che pur essendo uguali sia in entrata che in uscita sono tuttavia flussi finanziari che transitano per il bilancio) di rilevante ammontare. Le stesse relazioni, inoltre, non sono esaustive in ordine agli scostamenti tra previsioni e spese a consuntivo, soprattutto laddove si evidenziano notevoli «economie» sugli stanziamenti.

Un'analisi dettagliata, invece, avrebbe consentito di valutare i motivi di tali disallineamenti. Sempre con riferimento ai rendiconti, onorevoli Questori, in particolare ai relativi allegati, si nota che, per quanto attiene al Fondo di solidarietà tra i senatori, sono stati riportati i rendiconti del 2005 e del periodo 28 aprile-31 dicembre 2006, omettendo inspiegabilmente quello relativo al periodo 1° gennaio-27 aprile 2006, di pertinenza della XIV legislatura. Per quanto riguarda il Fondo di previdenza per il personale (Allegato G), il rendiconto 2006 riporta un bilancio del «Conto assicurativo individuale», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, un contributo degli iscritti, onorevole senatore Morando, di 530.808 euro ed un contributo del Fondo di 1.050.000 euro. del Fondo di 1.050.000 euro. Poiché è stato affermato, in sede di Consiglio di Presidenza, che esso si sarebbe autofinanziato, sarebbe interessante nella risposta capire in che modo, visto che il rapporto tra contributi degli iscritti e contributo del Fondo è di uno a due. In merito al preventivo 2007, si osserva in particolare che, proprio in ragione della contemporanea approvazione del rendiconto dell'esercizio anteriore, i raffronti tra le poste di bilancio avrebbero dovuto essere presentati con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente piuttosto che agli stanziamenti di preventivo, poiché solo così si avrebbe una percezione diretta e immediata del *trend* di spesa. Tutti i confronti proposti, invece, sono relativi al preventivo 2006.

per il quale è prevista una spesa di oltre 138 milioni di euro a fronte di un consuntivo 2006 di 128,9 milioni (cioè a dire con un incremento «reale», qualora la previsione venisse rispettata, del 7,12 per cento anziché del 3,58, come riportato nella tabella di pagina 29). Con riguardo alla tabella di raffronto con lo schema di bilancio, in uso fino allo scorso anno, sarebbe opportuno conoscere con quali criteri si è proceduto a tale applicazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, del Regolamento di contabilità approvato il 1° giugno 2006, che prevede che, ai fini di gestione, i capitoli siano suddivisi in articoli e che il Segretario generale - dice il Regolamento - determini la corrispondenza tra i capitoli, gli articoli, le aree omogenee di attività e gli uffici, in funzione di trasparenza e sistematicità. al comma 6, prevede, inoltre, che il bilancio preventivo sia corredato da un allegato - redatto in termini di competenza - nel quale siano indicati i contratti pluriennali.

L'elenco B), invece, riporta le somme impegnate ma non spese nel 2006 (i residui passivi) per un totale di 10,9 milioni di euro; si tratta di una cifra considerevole, tenuto conto delle dimensioni del bilancio del Senato.

poi dovranno parlare i senatori Questori, Comincioli, Nieddu e Thaler Ausserhofer; poi ci sono le dichiarazioni di voto: ne sono previste già tre, ma se ne è aggiunta - come avete sentito - una quarta. La sostanza della questione che voglio sottoporre a voi è questa: non è prevedibile la chiusura della seduta, sulla base dei tempi che abbiamo stabilito, prima delle ore 15,15. È evidente che non ci potrà essere nessuna interruzione e dovremo andare avanti. Allora, delle due l'una: o i colleghi si predispongono a rimanere sino alle ore 15,15 per votare il bilancio del Senato a quell'ora, oppure decidono, attraverso una forma di autocontrollo, di autodecisione, per carità, di non utilizzare interamente i venti minuti che sono loro concessi negli interventi, rivolgendo evidentemente il medesimo appello sia al relatore, che dovrà replicare, sia ai Questori. In questo modo potremmo forse concludere un po' prima:

perché non svolgo soltanto una valutazione ma forse possiamo anche ragionare su alcuni suggerimenti, sulle scelte possibili e future, per rafforzare la parte finale della relazione del senatore Morando. Infatti, *ictu oculi* oculi* (si veda la voce spesa riepilogo per titoli e categorie del documento numero 4) tutti i senatori potranno vedere dove sono le voci più rilevanti di spesa corrente strutturale.

che, presumibilmente, deciderà, delibererà, metterà mano ad una vasta riforma pensionistica dei nostri concittadini, e se anche così non fosse, comunque il problema, in sé, residuerebbe. Allora è del tutto evidente che, in un contesto pubblico dove tutto è trasparente a tutti e tutto va giustificato a tutti, è nostro dovere, sforzo, impegno intellettuale, impegno propositivo, offrire una qualche diagnosi e una qualche proposta di soluzione. Si dice che il vitalizio non è pensione normale: però si versano dei contributi;

Anche se non si tratta di pensione normale, certamente si versano i contributi e certamente va a premiare, a garantire un'importante funzione legislativa che si svolge per una parte della vita, e comunque un ruolo, una mansione che va giustificata,

Mi scuserà per l'imprecisione, ma il presidente del nostro Gruppo, Oskar Peterlini, se posso citarlo, mi raccontava di come la Regione a Statuto speciale Trentino-Alto Adige avesse, per i vitalizi dei consiglieri regionali, operato su una ristrutturazione dei contributi per mettere più in sicurezza l'intero sistema. Considerando il fatto che il vitalizio dei senatori e dei deputati si irradia su tutto il sistema dei vitalizi, ad esempio dei consiglieri regionali, e crea ormai una qualche riflessione pubblica di proporzionalità, io credo che se noi fossimo in grado di incidere, di giustificare e, come diceva il presidente Morando, di mettere in linea politica con il sistema pensionistico pubblico in evoluzione (già cambiato con l'introduzione del sistema contributivo), per questa parte, il sistema dei vitalizi parlamentari faremmo, come si dice, una cosa buona e giusta e daremmo anche dimostrazione di una buona pedagogia politica al Paese.

Siamo nell'epoca della comunicazione globale e quindi il tema della comunicazione interna ed esterna è centrale. In questo senso, devo anzitutto apprezzare la gestione e l'organizzazione del sito Internet del Senato, che è stato del resto riconosciuto a livello nazionale come uno dei siti istituzionali meglio organizzati. Se questo è vero, è altrettanto vero che risulta ad oggi del tutto incomprensibile l'assenza del Senato su Televideo RAI. La Camera dei deputati è presente in questo settore dell'informazione istituzionale con alcune pagine, devo dire, molto apprezzate, anche se, trattandosi di Televideo, abbastanza ristrette, ma efficacemente aggiornate: si tratta dell'ordine del giorno del lavori dell'Assemblea e degli ordini del giorno, continuamente aggiornati, dei lavori delle Commissioni, nonché di una sorta di estratto del resoconto sommario, che pressoché in tempo reale la Camera dei deputati colloca sulle reti principali della RAI, Rai Uno e Rai

c'era stato - sul Televideo della RAI, poiché ritengo sia un modo per essere apprezzati dai cittadini, da coloro almeno che sono interessati al funzionamento di un sistema che è tuttora bicamerale, quindi non si capisce perché sul Televideo vi debba essere lo spazio adeguato della Camera dei deputati e non quello del Senato. Un altro punto che riguarda la possibile integrazione e comunque il confronto con quanto avviene alla Camera dei deputati, ma che è più interno alla nostra organizzazione dei lavori, concerne la rassegna stampa quotidiana. La rassegna stampa della Camera dei deputati è, di fatto, duplice: esiste, come al Senato, una rassegna stampa cartacea

cartacea, potrebbero rappresentare uno spreco, ma che possono essere utili per i senatori e per quanti hanno accesso alla rassegna stampa. È vero che noi senatori possiamo accedere al sito Internet della Camera dei deputati, ma non si comprende perché un servizio di questo tipo non venga realizzato congiuntamente dai due rami del Parlamento o non sia comunque presente nelle stesse dimensioni anche nell'organizzazione del Senato.

Perché non realizzare tutti i giorni o, in questo caso, almeno nei principali giorni della settimana lavorativa, esclusi i festivi, la rassegna della stampa estera? Se c'è una collaborazione con il Ministero degli affari esteri, credo che questa non debba essere limitata ad un solo giorno alla settimana.

degli organi di informazione non italiani sia un modo più completo per mettere a disposizione dei senatori e di quanti hanno accesso ai siti del Senato una documentazione utile per il lavoro che si deve affrontare in un quadro di Europa unita e comunque di mondo globale sempre più interdipendente. Da ultimo avanzo un invito ad aggiornare al più presto, per quanto possibile, signori Questori, i sistemi operativi installati sui *personal computer* dei nostri uffici senatoriali. Sono al momento sistemi operativi abbastanza antiquati, tenendo conto naturalmente di come diventano subito

su Internet, per esempio audiovideo di incontri, manifestazioni o altre simili iniziative che si svolgono nel mondo e che sono accessibili sulla rete purché il sistema operativo ne consenta l'accesso.

prevalentemente alla scorsa gestione, tanto che si è avuta complessivamente una riduzione di uscite rispetto agli stanziamenti e alle entrate previste cento. Queste riduzioni e risparmi sono distribuiti su varie voci: relazioni esterne, trattamento di senatori ed ex senatori, personale in attività ed in quiescenza, attività di indagine, controllo e vigilanza, stampa degli atti parlamentari, comunicazione e documentazione, beni e servizi, trasferimenti ed altri, in cui non entro perché non aggiungerei niente a quanto è possibile leggere nel bilancio stesso. Bisogna notare invece che nei sei mesi successivi il risparmio è stato solo dei rimanenti 4,5 milioni di euro e che per il 2007

noi siamo una delle due Camere che producono leggi per il resto del Paese e, in quest'ultimo periodo, leggi finalizzate soprattutto a ridurre

prevedendo un incremento di spesa del 4 per cento, cioè il doppio di quella che dovrebbe essere l'inflazione prevedibile per l'anno in corso e, soprattutto, il doppio di quel 2 per cento la Casa delle Libertà aveva indicato come incremento massimo di tutto quello che è pubblico, statale, comunale, regionale o provinciale nel nostro Paese. Ecco, non vorrei che questo fosse un cattivo esempio che poi in qualche modo si ribaltasse su tutte le altre attività dello Stato aventi riflessi economici. In particolare, sono previsti alcuni incrementi di spesa,

forse per deformazione prima ancora che professionale direi territoriale, io sono abituato ad andare a vedere i dati che contano e che fanno subito cifra nei bilanci. Per cominciare, anche qui per sfatare qualche mito,

il costo complessivo dei senatori, quello cioè che nell'immaginario collettivo dovrebbe essere il costo del Senato, è pari a circa 160 milioni di euro (quindi circa al 32

Quindi, 1.100 dipendenti cominciano ad essere veramente tanti. Se pensiamo che alla Camera sono più di 2.000, che al Quirinale sono circa 1.200 e che alla Presidenza del Consiglio sono anche lì, più o meno, 1.100-1.300

che sono importanti anche in linea di principio. Se non cominciamo a ragionare dando un nome e un cognome ai problemi del Paese, difficilmente li risolveremo,

parte del meccanismo complessivo e quindi non ha una responsabilità diretta, sto parlando alle persone che gestiscono il complesso della macchina e che quindi su queste cose in qualche modo devono intervenire),

un ordine di grandezza. Vorrei invitare tutti, maggioranza e minoranza, opposizione presente e futura, maggioranza presente e futura, a fare delle riflessioni.

dopo; ciò che devo fare è indicare cosa serve per fare quello che devo fare. E se comincio ad avere parti di azienda (in questo caso, parti di Palazzo) che non servono più, non metto nessuno per strada, ma riconverto, riqualifico, non assumo per qualche anno, perché ho da ripiazzare le persone che ho già a disposizione. Questo significa fare un minimo di efficienza aziendale anche nella cosa pubblica. Ribadisco il concetto: 35 milioni di euro al mese di costo medio del personale è inaccettabile. La gente non si arrabbia perché si va in pensione o 60 o a 65 anni, cosa su cui magari si potrebbe anche ragionare: ma andate a dire al TG1 delle ore 20, mentre le famiglie italiane sono a casa a mangiare, che il dipendente medio della Camera o del Senato costa 35 milioni al mese al pubblico erario, e vedrete se il giorno dopo non c'è veramente la rivoluzione in piazza di 30 milioni di persone. persone. Sono cose su cui non si può fare finta di nulla. A fronte di questo, continuiamo a prevedere incrementi annuali che, anch'essi, sono fuori da ogni logica, da ogni situazione.

a cui abbiamo chiesto sacrifici, a cui avete chiesto di pagare più tasse, agli imprenditori che hanno le aziende che finiscono in pareggio ma devono pagare lo stesso 30.000, 40.000 o magari 60.000 euro di IRAP, anche se non hanno avuto nessun guadagno aziendale (perché è una legge che tassa il guadagno che non c'è, anzi, tassa l'occupazione), e se poi magari con questo sistema escono un pochino dallo studio di settore arriva subito il funzionario dell'Agenzia delle entrate accompagnato da due carabinieri a fargli le pulci nel bilancio e dargli magari altri 40.000, 50.000 o 60.000 euro di multa:

in questa situazione, soprattutto quando un'analisi critica di certi elementi non è minimamente accennata in tutte le relazioni che ho avuto modo

che paga le tasse e vota in un altro Paese, viene nel nostro Paese, dove non parla la lingua, non paga le tasse, finendo, come abbiamo visto in questa legislatura (ma poteva essere lo stesso dall'altra parte, non lo dico perché questa volta ha favorito voi), per decidere per 60 milioni di persone con cinque o sei voti di scarto.

dopo tre o quattro anni di nostra amministrazione, siamo arrivati a 70 dipendenti, senza licenziare nessuno, ma solo usando i trasferimenti, i pensionamenti, eccetera. Il Comune funzionava e funziona esattamente come prima, se non addirittura meglio. Ci sono tanti altri Comuni che, con 17.000 abitanti, hanno quattro o cinque volte i dipendenti che ci sono nel mio paese. La Regione Lombardia, con 10 milioni di abitanti, ha 2.300 dipendenti e la Regione Sicilia (parlo con rispetto per i siciliani presenti), con 5 milioni di abitanti, ne ha 26.000, cioè 12 volte di più, con metà degli abitanti. Andiamo poi sui giornali e in televisione a dire che il problema è il costo della cosa pubblica. Ma dov'è questo problema? C'è cosa pubblica e cosa pubblica, in Italia. C'è cosa pubblica che funziona, perché la gente ha il buonsenso di comportarsi come un buon padre di famiglia o come un qualunque imprenditore oculato che guarda soprattutto le uscite: riduce prima di tutto i costi e va poi a vedere le entrate. Ci sono, invece, persone che amministrano la cosa pubblica solo dal punto di vista delle entrate: tirano la somma a destra di quanto costa e vanno poi a chiedere le relative risorse ai cittadini sotto forma di tassazione. Questo non va bene come principio, ma soprattutto non risolve i problemi del Paese. Chiudo, per risparmiare qualche minuto.

Signor Presidente, ho ripresentato l'ordine del giorno G3, relativo alla questione dei collaboratori parlamentari, che l'anno scorso invece ritirai perché fu accolto come raccomandazione dai signori Questori. È certamente un po' mortificante, per il ruolo di un senatore, vedere che una questione posta correttamente in termini tecnici e formalmente non venga tenuta in debita attenzione e invece poi una trasmissione televisiva vista molto dai giovani - mi riferisco alle interviste de «Le Iene»

per cui preferisco, anche per *forma* *mentis*, non guardarmi indietro, ma guardare avanti. L'unica cosa che rammento è che nella dichiarazione di voto che feci l'anno scorso sulla materia dissi che fin quando questa tematica non fosse stata puntualmente risolta mi sarei astenuto sul bilancio

vorrei far rilevare al Presidente, e soprattutto al relatore Morando, alcuni aspetti. Non mi attardo su quelli già trattati dai colleghi o su altri, quali il personale, il trattamento pensionistico, gli immobili o la gestione, perché interverrà il mio collega Viespoli in proposito. So che si stanno facendo passi in avanti notevoli e quindi mi affido a lui quale rappresentante del Gruppo in questa

su alcune criticità che individuo innanzi tutto nella tempistica. Apprezzo quanto è stato fatto; ho letto con attenzione i bilanci e le rendicontazioni di quest'anno e li ho confrontati con quelli degli esercizi precedenti. Il rilievo critico è dovuto al fatto che io ho avuto questi documenti giovedì pomeriggio, per gentile concessione del presidente Morando che me li ha dati ancora in forma di bozza. Discutere oggi, a soli cinque giorni di distanza, compreso il fine settimana, appare un tantino prematuro perché non mi sembra che ci sia la sufficiente riflessione sui numeri e sui contenuti, quindi non è facile dare un contributo. È una personalissima opinione, che però sottopongo alla vostra attenzione per far sì che in futuro ci possa essere un maggior tempo disponibile tra il momento di presentazione degli atti nella forma ufficiale, e cioè dopo l'approvazione della Commissione presieduta dal senatore Morando,

perché un'Aula come questa, con al momento neanche una trentina di colleghi - stamattina ne ho contati 54 e spero di non avere sbagliato - per un documento così importante, che affronta gli oltre 500 milioni di euro di costo di questa struttura, forse meriterebbe un *quorum* per lo meno di un terzo dei senatori per rendere legittimo, consapevole e valido il voto. Anche questa è una banalissima proposta che sottopongo, non è un motivo di totale criticità, però certamente una partecipazione maggiore di tutti ci renderebbe più consapevoli. Io parlo *erga omnes*, verso tutti; poi ho difficoltà a guardarmi alle spalle perché, diversamente da te, non ho gli occhi anche da dietro. Passando a qualche altra considerazione critica,

e rilevo che anche l'estensione giurisdizionale dell'autodichia è un qualcosa che forse nella precedente legislatura non è stata sufficientemente considerata,

«chiarezza», «trasparenza», «lotta all'evasione fiscale e al lavoro nero» sono le parole più diffuse, però poi una certa coerenza non la intravedo in alcuni atti. Entrando più specificamente nel merito, credo che il bilancio che, ad esempio, non porta nulla dei bilanci dei Gruppi se non le somme trasferite, consente altre anomalie, per cui il lavoro nero che si è ipotizzato per i collaboratori parlamentari forse esiste anche all'interno dei Gruppi. Il fatto che non ci sia un regolamento per i criteri di approvazione dei bilanci dei Gruppi è un altro elemento, senatore Morando, di cui una persona sensibile come lei non può non tener conto e per il quale non può non favorire, insieme al Collegio dei Questori, qualche successiva regolamentazione, in modo tale da capire bene la famosa

nel limbo, non sarà mai affrontato da nessuno; ci dovremo accontentare di quello che ci viene detto senza aver nessuna prova certa del contrario. contrario. Concludo il mio intervento - perché vorrei rispettare almeno io l'impegno di ridurlo - annunciando che mi asterrò dal voto unicamente per quei princìpi richiamati già l'anno scorso, ma ho piena fiducia che il Consiglio di Presidenza e lo stesso ruolo del presidente Morando possano far sì che l'anno prossimo registreremo una tempistica più corretta

presentazione all'Aula (l'anno scorso come auspicio, quest'anno come risultato) di una situazione diversa per quanto riguarda il momento in cui il progetto di bilancio per l'anno in corso

avrà maggior significato se, oltre a poter svolgere tale dibattito prima che gli effetti trascritti e disposti nello stesso siano votati e deliberati, la discussione potrà avvenire in una valenza prospettica tal quale la stanno più volte auspicando

la prova che secondo noi si debba agire diversamente non è quello che si realizza negli enti locali, ma - come molti enti stanno variando la tipologia dell'assetto, della discussione e della formulazione del bilancio interno - è il fatto che nello Stato non ci sia chiaramente un bilancio di competenza economica, perché le risorse attinenti non sono rinvenienti da ricavi, ma solamente da manovre finanziarie. Auspichiamo infatti che il bilancio dello Stato di competenza giuridico-finanziaria e contemporaneamente di cassa e che, quindi, abbia una tipologia mista che ci possa consentire, non soltanto di verificare l'efficienza e la qualità della spesa, ma anche una progettazione e, a questo punto, di gratificare l'azione di amministrazione attraverso una ricerca di efficienza che può essere garantita scientificamente soltanto da un bilancio di tipo misto, cioè di cassa e di competenza giuridico-finanziaria. Dico questo

oggi, faccio un riferimento forte alla percezione esterna di quello che facciamo, tutti i giornali titolano: maggiori spese per il Senato. per il Senato. Quest'Aula voterà anche oggi favorevolmente il bilancio del Senato, che è teso a cercare di raggiungere una migliore efficienza e che ha registrato negli anni che vanno dal 2001 al 2007 una variazione annua sempre più

mentre ciò significa un grandissimo sforzo da parte nostra, non viene percepito all'esterno come il raggiungimento di un obiettivo. Dobbiamo discutere - questo è il il motivo che vorrei porre al centro del mio intervento - se esso rappresenta un sacrificio oppure una responsabilizzazione nell'azione amministrativa.

il sacrificio che viene operato da parte del Senato e da parte dei Questori sul contenimento delle spese, mentre non viene percepito all'esterno come un atto di grande responsabilità nella conduzione della cosa pubblica,

la differenza - ed è difficile che si capisca - tra privilegi e prerogative. Trattandosi di grandi difficoltà incontrate negli ultimi anni dagli italiani, dall'Italia tutta, abbiamo finito per considerare che le necessarie prerogative abbiano preso la configurazione di privilegi.

sia accompagnata da una comunicazione che faccia comprendere che il vitalizio nasce in tutti i Paesi per far sì che la politica non sia una prerogativa dei ricchi

di contribuire al fondo pensioni professionale. Ciò viene commisurato ai migliori dieci anni degli ultimi quindici anni di contribuzione e pertanto egli avrà completamente perso le contribuzioni precedenti. Pertanto, non si capisce bene come la sua attività parlamentare non debba essere garantita da un assegno vitalizio che faccia

dei sacrifici. Inseguiamo la necessità di diminuire le spese, per cui a un dato momento abbiamo certamente pensato che la biblioteca si dovesse unificare. È auspicabile che se la biblioteca si unifica, lo si fa anche per dimezzare le spese, perché è assurdo pensare che di due biblioteche, una della Camera e una del Senato, se ne faccia una ma che le spese rimangano le stesse. A questo punto, se il criterio deve essere quello

più efficiente, più compatibile con la necessità che si studi davvero, questo mi trova senz'altro d'accordo. Se si dice che bisogna diminuire il numero dei dipendenti del 5 per cento, se questo non diventa un atto di responsabilità, ma un sacrificio non sono d'accordo. Ripeto ancora, è utile pensare di diminuire la spesa del Senato quando tutti i giornali titolano «582 milioni per il Senato» e quando continuiamo a realizzare interventi rispetto al costo medio

ma soprattutto il completamento dei servizi e dei prodotti a supporto dell'attività parlamentare, del lavoro del senatore e della funzionalità degli Uffici devono essere il nostro obiettivo. Vediamo cosa significa questo

di rendere quest'Aula più coerente rispetto alla richiesta, di cercare di fare meglio il nostro dovere, di produrre leggi migliori, non già tentare di apparire all'esterno come salvatori della Patria portando ai limiti ultimi

colleghi, in seno al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 l'Assemblea è chiamata quest'anno ad esaminare due consuntivi, quello relativo all'esercizio 2005 e quello relativo al 2006. La novità, come è stato detto, è imputabile alla prima applicazione del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato dal Consiglio di Presidenza il 1° giugno 2006. Per la prima volta il rendiconto dell'anno finanziario appena trascorso, in questo caso il 2006, viene presentato all'approvazione insieme al progetto di bilancio di previsione per il nuovo esercizio 2007, mentre, come tutti sappiamo, prima della riforma il consuntivo veniva presentato all'Assemblea unitamente al bilancio di previsione del secondo anno successivo a quello cui il rendiconto si riferiva, perdendo così ogni carattere di attualità e di collegamento con il progetto di bilancio di previsione. È questo certamente un primo elemento positivo che si unisce al fatto che, con l'esame odierno da parte dell'Assemblea, l'*iter* di approvazione dei documenti di bilancio interno si conclude quasi nel primo trimestre dell'anno, nel sostanziale rispetto dei termini regolamentari. Come tutti sappiamo, la *mission* del progetto di bilancio viene individuata dal documento sulle linee guida dell'attività amministrativa, che, predisposto dal Presidente d'intesa con i senatori Questori, é stato già sottoposto all'esame del Consiglio di Presidenza lo scorso 6 dicembre 2006. Tale documento, all'interno di un macroquadro di contenimento della spesa, prevedeva alcune priorità: dalla possibilità di un'integrazione funzionale con l'altro ramo del Parlamento nella gestione dei servizi di documentazione e di informazione - si è parlato molto della Biblioteca alla destinazione di risorse prioritarie finalizzate, agli interventi per il rafforzamento dell'affidabilità e della sicurezza delle infrastrutture, dei servizi e prodotti a supporto dell'attività parlamentare e del lavoro del parlamentare, al miglioramento della sicurezza dei palazzi ed all'acquisizione, ove possibile, di nuovi spazi per concentrare la presenza dei parlamentari nei palazzi storici, decentrando i servizi amministrativi e di supporto; ancora, dalla politica del personale, con l'adozione di un piano quinquennale di reclutamento, che prevedeva anche ipotesi di razionalizzazione, fino allo studio di ipotesi di affidamento in *outsourcing* di alcune funzioni o servizi non strategici. Non sono in grado di verificare adesso se e come il progetto di bilancio riuscirà a garantire tali priorità, anche se qualche perplessità di contesto, in qualche modo, affiora e speriamo con il tempo possa essere fugata. Nel tentativo, però, di operare comunque una ricognizione, pur nella limitatezza dei limiti temporali, e a volere guardare, ad esempio, al dibattito che si è consumato lo scorso anno (era il 3 ottobre), ci sarebbe da prendere atto che alcune richieste sono rimaste sostanzialmente inevase o disattese. La proposta del collega Paravia, che viene ripresentata oggi, non ha avuto ancora una concreta attuazione, anche se sappiamo che è stata costituita una Commissione che valuterà la cosa; i posti fissi in Aula non sono stati ancora assegnati, pur avendo l'Assemblea espresso una precisa volontà in quell'occasione (l'approvazione dell'altro bilancio), respingendo l'ordine del giorno di segno opposto, presentato dal collega Malan e altri; ancora, rispetto alla richiesta avanzata dal presidente Calderoli alla fine della discussione, che era intesa a cercare di garantire servizi igienici più adeguati, dopo oltre sei mesi di lavoro, si è prodotto risultato che, a mio modesto avviso, è parziale, non è soddisfacente ed evidenzia danni accessori notevoli se è vero, com'è vero, che l'accesso all'Aula, a causa di un cedimento strutturale del solaio superiore, è diventato un corridoio di guerra con tubolari, transenne e divieti. Insomma, se dovessi ragionare soltanto sulla base di questi dati, dovrei riconoscere che non è un buon inizio. Ci sarebbe ancora tanto da dire, ma preferisco utilizzare il tempo residuo per illustrare i tre ordini del giorno che ho presentato. Non ho bisogno di far riferimento alla mia attività nell'organo di autodichia di primo grado per rilevare quanto l'ordinamento interno del Senato sia frutto di sedimentazioni successive, di esigenze nate in altre epoche, di normative spesso caotiche, confuse o scarsamente trasparenti. Basti solo ricordare che la previsione di giurisdizione nei confronti dei terzi, introdotta meno di due anni fa con una decisione del Consiglio di Presidenza, è stata oggetto di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, mentre non ha mai ricevuto analoga pubblicità il Regolamento che prevede la disciplina degli organi che quella giurisdizione debbono esercitare, con la conseguenza che i fruitori del servizio (ricorrenti interni ed esterni) non riescono a conoscere quali regole e quali preclusioni saranno applicabili concretamente alla controversia che li occupa. E questo purtroppo è assurdo. Voglio però soffermarmi preliminarmente, anche per illustrare l'ordine del giorno G5, su una peculiarità dell'ordinamento Senato, alla quale si è già fatto riferimento in altre sedi, anche di esame di precedenti bilanci interni. Il trattamento previdenziale, che per qualsiasi lavoratore pubblico o privato rappresenta un diritto costituzionale disciplinato da una normativa uniforme, negli organi costituzionali è normato con appositi atti interni che per il Senato coincidono con il Regolamento di quiescenza del personale. Rispetto a tale disciplina, le erogazioni previdenziali di provenienza dello Stato si configurano come sotto dettatura, quasi che la tutela della posizione costituzionale dell'organo determini automaticamente la intangibilità delle pensioni dei suoi dipendenti. Se stessimo ancora all'epoca dei conflitti fra Real Casa e Camera elettiva capirei, ma ora è abbastanza difficile. Non soltanto tutto ciò produce discipline differenziate fra gli organi costituzionali, ma assoggetta al classico *dictum principis* quello che per tutti i dipendenti pubblici è, e deve essere, invece, un diritto costituzionale. Potrebbe apparire conveniente, ed in effetti lo è stato finora, avere una normativa di nicchia, al riparo della posizione costituzionale del datore di lavoro, ma ciò comporta delle vere e proprie aberrazioni, come quella, più volte denunciata da ultimo anche dal relatore Morando, che immagina però soluzioni diverse, relativa alla carenza di una disciplina pensionistica per i dipendenti assunti dopo il 1998. Inoltre, come spiegato dalla Commissione contenziosa si devono riscontrare solidi motivi di ordine pubblico, di ordine giuridico inerenti allo *status* che alle Camere compete per espressa previsione costituzionale per impedire l'applicabilità della regolamentazione ai dipendenti di un autonomo potere dello Stato. Tanto sullo sfondo del principio secondo il quale solo in via di eccezione si può negare l'applicabilità ai dipendenti delle Amministrazioni parlamentari del trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, e faccio riferimento alla decisione n. 282 del 2006. Invocando la giurisprudenza amministrativa più evoluta - che distingue la qualificazione giuridica del rapporto di servizio dalla riconducibilità dell'Amministrazione ad un potere dello Stato diverso dall'Esecutivo la Commissione contenziosa ha già ritenuto estensibile all'Amministrazione del Senato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esattamente come per gli appartenenti all'ordine giudiziario. È allora preferibile una stabilizzazione anche normativa del rapporto previdenziale, non solo per i giovani dipendenti ma per tutti. L'opportuno riconoscimento della specificità degli organi costituzionali, posti nel cuore dello Stato, merita uno scorporamento dalla platea generalizzata degli enti previdenziali dei dipendenti pubblici. Ma ciò si può conseguire razionalmente: con l'attuale sistema, la dotazione ordinaria annuale va a coprire le spese per il trattamento di quiescenza nella loro integrità. Occorrerebbe invece che, su un piano di assoluta parità, gli organi costituzionali (od a rilevanza costituzionale che versano nella medesima condizione del Senato) costituiscano un Fondo di previdenza unico, la cui disciplina sia concordata in maniera unitaria e la cui gestione sia affidata ad un consiglio di amministrazione in cui ciascun organo detenga un solo voto. Il costo iniziale, per tale fondo, dovrebbe essere quantificato previ contatti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministero dell'economia e delle finanze: la fiscalità generale potrebbe assumersene in parte l'onere, che sarebbe comunque meno ingente proprio con una platea di interessati più ampia del solo del solo Senato; ma, soprattutto, tale onere sarebbe trasparente, mentre finora si è versato in uno stato di permanente opacità, in cui i costi previdenziali del personale erano «nascosti» nelle pieghe di apposite voci di bilancio interno. Onorevoli colleghi, so di enunciare verità sgradite a taluno, ma un profilo di indipendenza di giudizio, nell'affrontare le complesse questioni dell'organizzazione interna delle Camere, è consigliabile; esso è addirittura richiesto dalla sentenza 6 maggio 1985, n. 154, della Corte costituzionale quando si versa in ambito giurisdizionale. Ecco perché (e faccio riferimento all'ordine del giorno G4, firmato insieme al collega Calvi, relativo agli organi di autodichia) la posizione di indipendenza del giudice rispetto all'Amministrazione necessita di essere garantita con appositi conferimenti: la filiera gerarchica rappresenta oggettivamente un'anomalia, anche quando è filtrata con sagacia e grande professionalità dal personale di segreteria di cui disponiamo. La possibilità di attivare rapporti consulenziali e di segreteria particolare, avanzata dai miei predecessori nella Presidenza della Commissione contenziosa, non va letta come una pur doverosa salvaguardia della *par condicio* con gli altri organi collegiali del Senato, ma come una autentica opportunità di offrire alla "necessaria indipendenza" ed alla qualità della produzione degli organi il supporto di esperienze professionali - nel campo del diritto - almeno pari alla bisogna. Perché a fronte di ricorsi sempre più complessi, redatti da studi professionali esterni, sempre sintonizzati sui più recenti sviluppi di giurisprudenza in materia appaltistica, ed a fronte dell'elaborazione difensiva dell'Amministrazione (che attiva consulenze da anni in questo settore, ricorrendo ad autorevoli figure della giurisdizione amministrativa), mi pare doveroso che la Commissione contenziosa ed il Consiglio di garanzia si attrezzino per offrire all'organo decisorio un supporto conoscitivo adeguato. Non mi pare che il Collegio dei senatori Questori abbia colto l'importanza di questa richiesta, che mira a garantire l'indipendenza e la professionalità degli organi e quindi di riflesso la credibilità dell'Istituzione Senato, avendone più volte rinviata la trattazione per un presunto approfondimento, quasi utilizzando una logica paramercantile. È però vero che altre priorità ricevono attenzione: è per offrire un contributo, per indirizzare al meglio tale attenzione, che ho proposto il terzo ordine del giorno (il G6). Con esso si mira a ricondurre in *bonus* anche se il mio ragionamento è abbastanza astratto - la politica delle spese per le pubblicazioni del Senato - e come tali intendo sia quelle prodotte, che quelle acquistate, che quelle distribuite un'accezione che potrebbe essere considerata retriva e superata delle spese di rappresentanza. Non ho bisogno di ricordare come la sezione giurisdizionale per la Regione Calabria con la sentenza n. 109 del 2006 abbia escluso che l'immunità funzionale di organi elettivi a rilevanza costituzionale copra l'esorbitanza rispetto alle finalità tipiche del potere di auto-organizzazione. Basti pensare che i principi ispiratori della destinazione dei fondi pubblici alle spese di rappresentanza sono: la concreta ed obiettiva esigenza di un ente, in rapporto ai propri fini istituzionali, di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei; l'idoneità dell'attività di rappresentanza a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'amministrazione, dimostrando il nesso temporale e/o modale tra spesa e circostanze che l'hanno originata; l'esclusione - sottolineo «l'esclusione» - di ogni forma di rappresentatività all'interno all'interno dell'ente, tra i suoi organi, ovvero tra essi ed i propri dipendenti o altre persone fisiche istituzionalmente operanti nel suo ambito; e la preventiva definizione, in termini essenziali, dell'esigenza di rappresentatività dell'ente, tramite atti regolamentari o atti amministrativi generali. Anche su tutto ciò sarebbe assai opportuno ricevere dal Collegio dei Senatori Questori le opportune delucidazioni, che coprano sia l'attività sin qui svolta, sia quella che si intende mettere in campo per il futuro, per verificare se il Senato sia effettivamente sintonizzato con quei principi di buona amministrazione prescritti dalla legge che valgono per tutti, senza eccezione alcuna.

non servono assolutamente a niente. È l'invio, per esempio, della *Gazzetta Ufficiale* che 1.000 parlamentari ricevono circa 365 giorni l'anno. So che è una competenza incrociata perché ho chiesto che non mi venissero più inviate: non si capisce se la competenza è del

Si fanno delle pubblicazioni oggi - perché così è sempre stato - del tutto anacronistiche. Pensiamo ormai che le banche dati informatiche sono lo strumento più utilizzato, il più pratico e meno costoso, oltre al resto, a cui tutti si rivolgono.

Suggerirei al Senato, nella veste del Presidente, e ai senatori Questori magari di scrivere una lettera ai senatori, visto che questa è l'unica loro competenza in tal senso, se intendano ancora ricevere a domicilio questi documenti.

Non siamo dei draconiani, non vorremmo vedere tutti appiedati, tutti con il saio; non siamo dei Savonarola. Però, se esiste un certo decoro istituzionale per cui è necessario offrire un minimo di servizio e di rappresentanza

sul servizio di autonoleggio. Questo non tocca più il Senato ma la Presidenza della Repubblica: le automobili di servizio sono 40. La Casa Bianca, un'altra struttura presidenziale, ha soltanto 5 automobili di servizio. Questo la dice lunga su come noi andiamo avanti con un sistema senza mai

Presidente, sarò molto breve, anche perché per conto dell'UDC ha parlato il collega Eufemi e non devo aggiungere molte considerazioni. Ad una però tengo particolarmente: per circostanze che onestamente non so basate su cosa, vi è nell'opinione pubblica una convinzione

allora formalmente ai senatori Questori che su tale questione facciano una pubblica conferenza stampa, portando i testi vigenti, dai quali risulta in modo tassativo che non esiste alcun convivente al quale spetti alcun diritto di alcunché. Perché l'opinione pubblica, diceva giustamente il collega Galli, non tollera i privilegi per i parlamentari, se non sono giustificati da questioni di ordine costituzionale, e in materia di conviventi non vi sarebbe alcuna ragione al mondo. Poiché allora nessuna delle normative vigenti

vigenti alla mano, non con parole o chiacchiere, che non esiste alcuna reversibilità a favore di alcun convivente. Questo va detto, perché non possiamo tollerare più che esista un'opinione pubblica disinformata sulla natura dei nostri comportamenti economici. [**Presidenza secondo punto riguarda sostanzialmente la natura dell'istituzione Senato. Io chiedo per quale ragione, ora che il Senato è diventato molto più rilevante anche dal punto di vista politico, su Televideo

terzo luogo, noto con qualche preoccupazione che molti giovani funzionari del Senato attendono decisioni che riguardano le nomine, che mi dicono non sono state fatte da più di un anno.

come è possibile che il Senato, che fa cose molto rimediate, possa avere bisogno di una quantità così enorme di persone? Questo è un problema specifico, occorre capire dove vengono collocate queste persone; ma perché non sono state fatte nomine? Se invece queste nomine sono state fatte, allora chiedo scusa per aver detto una cosa non vera. Sulla prima questione, ripeto e concludo, è fondamentale che il Senato della Repubblica, nella persona del Presidente - ma forse sarebbe eccessivo - o certamente dei colleghi senatori Questori, dica che non esiste alcuna norma vigente che preveda il convivente quale titolare dei diritti dei dei senatori, perché non è vero e occorre che lo si dica ufficialmente. Non è vero. Occorre che questo venga detto con l'ufficialità che i senatori Questori possono avere. Noi come Gruppi lo faremo, possiamo farlo, ma possiamo anche non essere creduti; i senatori Questori

hanno lamentato che io, addirittura per pochi secondi, abbia abbandonato l'Aula e non abbia ascoltato gli interventi. Era una telefonata cui non potevo rispondere: «Sono impegnato»; mi limito a dire questo e mi scuso con il collega

molto schematicamente riassumo su alcuni problemi che mi sono sembrati sollevati con particolare insistenza e con un orientamento che mi è parso unanime. Primo problema: l'obiettivo di riduzione del personale del 5 per cento. È stata posta esplicitamente la questione: in meno rispetto a che cosa? L'orientamento che io ho riconfermato nella mia relazione (che ha incontrato il favore, ho visto, non solo del senatore Grillo ma anche dei colleghi della Lega) è l'esigenza di precisare che quando si parla di riduzioni del personale e ci si dà un obiettivo si deve parlare degli organici di fatto e non di quelli di diritto, perché gli organici di diritto sono, anche per il Senato (mi sono dato cura di controllare), molto al di sopra del numero dei dipendenti attualmente in servizio al Senato.

dobbiamo esplicitamente modificare l'orientamento del Consiglio di Presidenza e precisare che si tratta del 5 per cento in meno rispetto agli organici ad una certa data. Se vogliamo dire che è alla data di oggi, diciamo che è la data di oggi, ma il riferimento al 5 per cento in meno rispetto ad una pianta organica che è di 200 addetti superiore rispetto al numero degli attuali dipendenti del Senato è un obiettivo patentemente non credibile, non si può considerare, considerare, secondo me, come un obiettivo che abbia una qualche credibilità. Sono d'accordo con il senatore Ferrara: quando ci diamo obiettivi di questo tipo non lo facciamo per rispondere ad una campagna demagogica nei confronti delle spese degli organi costituzionali: lo facciamo in funzione di obiettivi di qualificazione del nostro lavoro e di accrescimento della credibilità politica nel rapporto tra il Senato e l'opinione pubblica, i cittadini italiani. Se abbiamo un orientamento per il Senato può svolgere bene la sua attività e questa attività può essere svolta addirittura meglio anche attraverso una riduzione del numero dei suoi dipendenti, naturalmente procedendo ad una ristrutturazione, credo si debba essere fedeli a quell'obiettivo enunciandolo in modo credibile, e in modo credibile deve essere enunciato con rapporto agli organici di fatto. Secondo l'intercameralità dei servizi di documentazione. Ne ho parlato nella relazione, apprezzando i passi avanti che sono stati compiuti in quest'ultima fase: la Biblioteca, le scelte per il Servizio del bilancio. Mi è parso di cogliere degli orientamenti favorevoli molto diffusi da parte di tutti i colleghi che sono intervenuti. Vorrei dire, anche qui interloquendo, se mi si consente, con il senatore Ferrara, Ferrara, che io stesso nella relazione, quando con riferimento al Servizio del bilancio ho parlato di unificazione dei Servizi di bilancio di Camera e Senato nel Servizio di bilancio del Parlamento, ho detto che naturalmente all'interno di quel Servizio unificato dovrebbero agire due sezioni distinte che svolgano il lavoro di esame della corretta copertura delle leggi seguendo l'attività legislativa della Camera e del Senato. Finché esiste il bicameralismo perfetto potrebbe esserci il Servizio unificato per le attività di analisi e di documentazione sugli andamenti di finanza pubblica, risultando chiaro che all'interno di quel Servizio ci dovrebbero essere due sezioni assolutamente separate. Ovvero, si può del Servizio unificato del Parlamento per l'analisi degli andamenti di finanza pubblica, che poi ha al proprio interno due Servizi del bilancio, uno della Camera e uno del Senato, che svolgono l'attività a supporto dell'attività legislativa sul tema specifico delle coperture. Se così è, quindi se siamo tutti d'accordo, benissimo, su questo punto della intercameralità acceleriamo rispetto ai passi già molto importanti, al ritmo che i passi hanno assunto nel corso di quest'ultima fase. Diamoci l'obiettivo, colleghi Questori, signor Presidente, di avere per febbraio, quando discuteremo il prossimo bilancio di previsione, risultati importanti, per esempio sul terreno, non ancora dell'unificazione, ma del rafforzamento e dell'integrazione dei due Servizi del bilancio di Camera e Senato, con risultati già tangibili. A me sembra che questo sarebbe un passo importante nella direzione giusta.

Non c'è dubbio che questo è un elemento negativo. Io tale lo considero. So benissimo che per tutti i lavoratori il tasso di inflazione programmata viene assunto a base dei rinnovi contrattuali e che poi ulteriori aumenti sono possibili in rapporto alla verifica degli aumenti di produttività. Mi chiedo francamente perché sistematicamente al Senato, ma anche alla Camera e in altri organi costituzionali, non si segua esattamente questo stesso criterio

dei dipendenti del Senato si possa assumere questo riferimento: l'intervento di aumento deve essere quello relativo al tasso di inflazione programmata e al di sopra di quel livello si va in rapporto al conseguimento di precisi obiettivi di produttività. Se non assumiamo questo schema di riferimento continueremo a far danni perché non c'è dubbio che consentire sistematici aumenti al di sopra del tasso di inflazione programmata, nel momento in cui il Paese assume per i rinnovi contrattuali di tutti i lavoratori italiani (privati, pubblici) quel riferimento, è qualcosa che appare come un ingiustificato privilegio. Secondo me lo appare semplicemente perché lo è. quarto punto, quello dei trattamenti vitalizi per gli ex parlamentari, ha ragione il senatore Grillo. Credevo di averlo detto nella relazione, ma se non sono stato chiaro lo preciso meglio.

all'opinione pubblica sopra le innovazioni che questo sistema ha conosciuto, in particolare nel 1997, anzitutto per chiarire ciò che si dice che è, ma

D'Onofrio ha chiesto di precisare. Io non sono Presidente del Senato, non sono un Questore, ma sono in grado, avendo studiato il sistema, di escludere che ci sia questa previsione che - sottolineo - persino alcuni colleghi senatori pensano invece sussistere. Evidentemente c'è un equivoco che riguarda la reversibilità (che non c'è per il convivente), rispetto al fatto che le assicurazioni sulla vita, al pari di qualsiasi assicurazione, indicano il beneficiario nella persona indicata dal soggetto contraente l'assicurazione. Cosa c'entri però questo con la reversibilità del vitalizio è assolutamente imperscrutabile. Qualsiasi assicurazione sulla vita, al momento della stipula, prevede che colui che la stipula indichi il beneficiario in caso di premorienza. Confondere Confondere una cosa con l'altra è privo di senso per definizione. Noi dobbiamo dire bene quel che non c'è (ho appena fatto un esempio, riferendomi all'intervento del senatore D'Onofrio) e dobbiamo dire decisamente meglio quel che c'è,

1998, in sede di finanziaria (lo ricordo perché fui io a presentare quell'emendamento) proponemmo che i lavoratori dipendenti senatori, che sono iscritti a forme di previdenza pubblica, paghino loro, a carico del proprio reddito, la quota dell'8 per cento di aliquota contributiva, trasformando l'aliquota da figurativa in reale. Abbiamo quindi introdotto un ulteriore elemento di aggiustamento del sistema, nel senso di mettere a carico del lavoratore ciò che a suo carico deve rimanere. deve rimanere. A questo proposito va detto, signor Presidente, che nella fase di transizione si pone - cambiato quel che c'è da cambiare - il problema che si pone per il sistema previdenziale nel suo complesso. Perfetta la legge Dini a regime, nella fase di transizione si pongono una serie di problemi. La fase di transizione a regime definito per i vitalizi nel 1997 è, signor Presidente, secondo me, troppo lunga e quindi bisognerebbe realizzare un intervento su quel versante perché - lo dice un senatore che è alla quarta legislatura - non c'è dubbio che i senatori di maggiore anzianità di anzianità di legislature già effettuate sono in larga misura sottratti a quelle norme e ciò determina la possibilità di continuare in una campagna che sottovaluta il rilievo delle decisioni assunte nel 1997, nel 1997, che hanno modificato soprattutto l'età di accesso in modo determinante nel senso che ha indicato il senatore Grillo e che io non ho ragione di riprendere adesso. Bisogna però, secondo me, per mettere in relazione bene il sistema dei vitalizi con l'opinione pubblica italiana, realizzare un ulteriore intervento. Non sono io che devo realizzarlo, ma segnalo un problema

esageratamente alte, troppo premianti. Bisogna assolutamente aumentare, secondo me, quell'aliquota contributiva. In secondo luogo, abbiamo un regime del cumulo - ne ha accennato la senatrice Negri - troppo favorevole,

la situazione sta diventando, per alcuni aspetti, addirittura paradossale, secondo me, e comunque segnalo il problema perché mi sembra che ci sia. Ancora, il regime del riscatto, ovvero regime del riscatto, ovvero le somme che si devono versare quando i contributi non abbiano completato il periodo di riferimento e quindi quanto si paghi per acquisire il diritto avendo avuto la contribuzione di accedere alla prestazione. Non c'è dubbio che c'è oggi un calcolo delle quantità di riscatto che sono troppo generose rispetto ai soggetti interessati. Non capisco perché non si dovrebbe adeguare questo livello del riscatto alle prestazioni. Infine, non vi è dubbio che ci sono alcuni aspetti, oltre a quello di cui parlava il collega D'Onofrio, riguardo al regime di reversibilità penso per esempio all'assoluta indifferenza del reddito del soggetto superstite, assolutamente oggi non influente nel determinare il regime di reversibilità - indubbiamente troppo vantaggiosi rispetto al regime della reversibilità previsto per il resto del Paese. Vede, signor Presidente, noi possiamo anche dire che di tutto ciò si occupano i demagoghi, ma non è vero. Di tutto ciò devono occuparsi le persone serie che lavorano qua dentro e che sono la stragrande maggioranza, perché noi abbiamo un problema prima di tutto, che è quello del rapporto positivo con il Paese. Ho fatto nel corso degli ultimi 200 giorni giorni forse un centinaio di assemblee sulla legge finanziaria, assemblee popolari, riunioni nelle quali viene gente prevalentemente orientata nella stessa direzione in cui sono orientato io (sappiamo che parliamo ai nostri, come si dice, in queste assemblee); prego i colleghi di considerare - ma sarà esperienza comune - che appena si affronta il tema della necessaria politica di stabilizzazione, della necessaria politica di risanamento, il tema dei nostri trattamenti, del trattamento previdenziale dei dipendenti degli organi costituzionali, dei vitalizi dei parlamentari, viene proposto non da parte di chi fa qualunquismo, non da parte di chi vuole per forza ricercare la polemica, ma da parte di chi cerca un equilibrio, di chi è pronto a ragionare delle esigenze di intervento ulteriore sul sistema previdenziale però vuole vedere una coerenza complessiva del nostro atteggiamento. Penso che ne va della nostra credibilità e anche della nostra forza politica, non di questa o quella parte, ma

colleghi, prima di entrare nel merito degli interventi sviluppati in questo dibattito e dei contenuti degli ordini del giorno presentati dai colleghi mi sia consentito un saluto e un apprezzamento, a nome del collegio dei senatori Questori, al Segretario generale, ai vertici dell'Amministrazione e a tutto il personale, che quotidianamente mettono a disposizione dell'attività parlamentare e dei senatori la più leale collaborazione ed un patrimonio di professionalità e di dedizione invidiatoci da più parti. Mi soffermo in primo luogo sugli interventi del senatore Morando, indugiando brevemente su due questioni riguardanti direttamente la struttura del bilancio di previsione. È stato ripreso il tema del bilancio di competenza quale strumento di informazione e di elaborazione per grandi aggregati di spesa e di entrata in grado di dare il senso del carattere pluriennale degli impegni. Non posso in proposito che richiamare le considerazioni già espresse in altra occasione, cioè in occasione del precedente esame del bilancio e anche nei giorni scorsi nella Conferenza dei Presidenti di Commissione, limitandomi a ribadire che le giuste esigenze informative poste dal presidente Morando, come ad esempio quelle relative alle prevedibili evoluzioni della futura spesa previdenziale, non possono essere certamente soddisfatte attraverso i dati di un bilancio di competenza, ma devono essere oggetto di specifiche indagini prospettiche

confronto fra l'Amministrazione e i sindacati per i temi relativi alla previdenza del personale. Si tratta, dunque, di informazioni di carattere necessariamente aggiuntivo che possono trovare adeguato riscontro in specifici e separati documenti di programmazione economica e finanziaria. È un dato di fatto che emerge anche dall'analisi comparata di altri bilanci di competenza, come ad esempio quello della Camera dei deputati. Senza alcun intento polemico, al momento ritengo che le informazioni che può dare un bilancio di competenza finanziario di carattere annuale siano assolutamente soddisfatte dagli allegati al documento di bilancio e in particolare dall'elencazione dei residui registrati alla chiusura del precedente esercizio, dal quadro analitico degli impegni contrattuali che gravano sul corrente e sui prossimi esercizi e, infine, dal bilancio triennale. In ogni caso, le riflessioni sul punto andranno approfondite procedendo, tuttavia, con cautela nel continuo aggiornamento delle strutture e dei documenti contabili, valutando in particolare se le inevitabili complicazioni amministrative, come quelle derivanti da una formale gestione dei residui, siano funzionali ad un effettivo miglioramento della significatività dei bilanci e se non si rischi, invece, di accrescere quelle attività e le connesse risorse di spesa e professionali di autoamministrazione che si intendono ridurre a favore alla attività di *front office* e di diretto supporto all'attività legislativa e di sindacato del Governo, prospettata in un altro punto della relazione, correttamente di focalizzare le risorse e le attività verso il cosiddetto *core business* dell'istituzione Senato. Senato. Quanto ai rilievi sulla consistenza dei fondi di riserva rinvio alla relazione al progetto di bilancio e richiamo in questa sede quanto ho già detto detto nel corso della riunione dei Presidenti delle Commissioni permanenti. In una struttura come quella delineata nel nostro bilancio, dove gli appostamenti sono la più diretta e rigorosa rappresentazione degli impegni e dei progetti già definiti, i fondi di riserva rappresentano l'unica risorsa nella nostra disponibilità per affrontare una serie di questioni non ancora definite, piuttosto rilevanti e incombenti, come quella ad esempio dell'eventuale finanziamento a nostro carico degli interventi di ristrutturazione già iniziati presso il complesso di Santa Maria in Aquiro e dell'immobile di largo Toniolo, ove non dovessero sbloccarsi i finanziamenti a tal fine previsti dal bilancio dello Stato per il Provveditorato per le opere pubbliche. Il fondo di riserva è l'unica risorsa disponibile anche per far fronte a situazioni impreviste come, ad esempio, l'intervento resosi necessario per il rafforzamento del solaio sovrastante le sale contigue all'Aula, o qualsiasi evenienza imprevista ed imprevedibile dovesse verificarsi. Essi pertanto non devono apparire eccessivi, quanto piuttosto - lo ribadisco - l'espressione di un atteggiamento prudenziale per garantirci un ragionevole spazio di autonomia finanziaria e la possibilità di affrontare situazioni impreviste e decisioni operative con efficacia ed immediatezza. Di maggiore spessore, e pertanto meritevoli di un più ampio approfondimento, sono le questioni riguardanti il trattamento vitalizio degli ex senatori, da una parte, e la politica del personale dipendente, dall'altra. È stato espressamente ricordato che gli assegni vitalizi degli ex parlamentari non sono pensioni, da un punto di vista tecnico, ma sono percepiti dall'opinione pubblica come tali. Da tale premessa sono derivate una serie di considerazioni che sarebbero fondate ove parlassimo di un sistema previdenziale: ad esempio, quando si considera precaria la sostenibilità finanziaria del monte assegni vitalizi per l'asserito squilibrio tra contributi e prestazioni. In realtà, i vitalizi degli ex parlamentari hanno ben poco in comune con i trattamenti pensionistici. Al di là delle ben note differenze tecniche e giuridiche, qui mi preme sottolineare che una cosa è un trattamento di quiescenza che conclude naturalmente una vita lavorativa con il suo sviluppo di carriera ovvero di attività professionale, altra cosa è un trattamento, quale appunto il nostro vitalizio, che è teso a garantire che è teso a garantire un tenore di vita almeno decoroso a chi ha dedicato una parte considerevole della propria esistenza all'attività politica e legislativa, compensando in tal modo gli innumerevoli sacrifici, inclusa la rinuncia a prospettive di impegno, di successo e di soddisfazioni professionali. Passando all'esame dei profili tecnici, osservo che vi sono enormi differenze tra i trattamenti pensionistici e i vitalizi degli ex parlamentari. Infatti, in un sistema previdenziale la quota di gran lunga più rilevante dei contributi è a carico del datore di lavoro. Nel nostro caso tale quota manca del tutto, poiché il Senato non ha un rapporto con il parlamentare rapportabile a quello di datore di lavoro. Inoltre, l'intero ammontare dei contributi, ossia quelli pagati dal lavoratore più quelli pagati dal datore di lavoro, dovrebbe essere costantemente rivalutato in base ad un congruo tasso di capitalizzazione. Ciò non toglie che si debbano approfondire alcuni punti specifici cui ha fatto cenno il presidente Morando e poi il senatore Grillo, a cominciare dal loro riconoscimento del rilievo avuto dalla riforma degli assegni vitalizi già compiuta nella XIII legislatura, specie per quello che è stato chiamato il drastico innalzamento dell'età anagrafica di accesso alle prestazioni. Concordo su questo giudizio poiché è stato importante, sia sotto il profilo politico, sia per la sostenibilità finanziaria, avere innalzato la soglia di accesso all'età di 65 anni, riducibili fine alla soglia di 60 per chi abbia almeno dieci anni di contributi. Peraltro, anche questo intervento riformatore può essere rafforzato, soprattutto nell'ipotesi in cui una riforma pensionistica generale dovesse progressivamente elevare la soglia per la pensione di anzianità al di sopra dei 60 anni. Non vi sono tabù da questo punto di vista che non si possano discutere, ed alcune ipotesi sono stati richiamate in diversi interventi; ma eventuali ulteriori riforme vanno rese coerenti con un sistema normativo che disciplina lo *status* economico dell'ex parlamentare nel suo complesso e non può che essere uniforme per il Senato e per la Camera. Né si può dimenticare che uno *status* simile è previsto anche per i parlamentari europei e per i consiglieri regionali alla cessazione del mandato. condivido pienamente l'esigenza, recentemente affermata dal presidente Bertinotti, di salvaguardare i diritti acquisiti dai parlamentari che hanno già versato contributi per vari anni sulla base della normativa vigente. Un'eventuale riforma dovrebbe perciò andare a regime a partire dalla prossima legislatura, così com'è stato per le riforme precedenti che hanno rinviato a quelle successive l'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tale questione - concludo con una riflessione del tutto personale - rinvia ad una discussione più generale sui costi della politica da tempo aperta nel Paese,

Negare o fornire in modo inadeguato risorse alla politica o presentare queste alla stregua di una «grassazione», come pure è avvenuto in alcune campagne di stampa (non dobbiamo nasconderlo), significa colpire al cuore la democrazia, perché equivale a non riconoscere o a ledere il principio dell'uguaglianza politica dei cittadini, riproponendo senza dichiararlo ma in sostanza la discriminante di censo per la partecipazione alla vita pubblica: in altre parole, l'idea per la quale chi è più ricco avrà maggiori possibilità di partecipare alla vita pubblica e dunque decidere per tutti; negare mezzi e risorse alla politica vuol dire lasciare spazio a gruppi e persone dotati di una forte disponibilità finanziaria. Il senatore Manzella, nel suo intervento, ha citato lo Statuto albertino e sappiamo come il Senato del Regno venisse composto, chi potesse accedervi ed in quali forme tale accesso fosse consentito a taluni e non ad altri, cioè alla maggior parte dei cittadini italiani dell'epoca. Tutto ciò, dunque, dovrebbe allarmare ogni sincero democratico. Perché, allora, continua questa forte campagna che investe determinati soggetti, siano essi istituzioni, partiti o parlamentari e che si esprime contro le risorse pubbliche a sostegno della politica? La risposta a tale interrogativo è affidata a ciascuno di noi. Personalmente ritengo non sarà un bel giorno quello nel quale alla limitazione della libera espressione della rappresentanza democratica degli interessi farà seguito magari la forza di potentati economici o di censo; non sarà un bel giorno perché saranno indeboliti la democrazia, il libero confronto e la competizione, falsandone in partenza gli esiti. A proposito di informazioni su queste materie, devo sottolineare che il Collegio dei Questori, la Presidenza del Senato ed il presidente Marini hanno sempre fornito agli organi di stampa tutte le informazioni richieste, oltre a quelle che sono già di pubblica evidenza sul sito Internet del Senato, dove si può rinvenire tutto quel che riguarda tale materia. Oltre a ciò, a richiesta di diversi organi di stampa, fatto salvo il diritto di *privacy*, sono state fornite tutte le ulteriori informazioni. Quindi, non c'è nulla da nascondere, ma si deve affrontare un limpido confronto pubblico e democratico su queste materie perché i termini della questione vanno ben al di là della mercede di una prestazione lavorativa e riguardano lo *status* e le caratteristiche della nostra democrazia, della sua rappresentanza e del suo e del suo modo di essere. Quanto al sistema previdenziale del personale, il Presidente del Senato ha avviato personalmente le trattative con le organizzazioni sindacali dei dipendenti sul tema pensionistico con una riunione tenutasi il 19 dicembre 2006. A tale riunione, (avvenuta poco dopo l'esame del precedente bilancio nel quale la questione era stata proposta), nell'ambito della quale è stata illustrata una proposta di modifica alla disciplina oggi vigente, ne sono seguite molte altre nell'arco degli ultimi tre mesi e mezzo, sia a livello di rappresentanza permanente per le questioni del personale (l'ultima si è tenuta giovedì scorso e vi abbiamo partecipato direttamente), sia a livello di tavolo tecnico-amministrativo. Trattandosi di una problematica complessa e che coinvolge un aspetto molto importante del rapporto di lavoro, peraltro aperto e irrisolto dal 1998, è comprensibile che la trattativa non sia ancora potuta potuta giungere nell'arco di poche settimane ad una conclusione. Come annunciato nel corso di questa seduta dal presidente Marini, è stato già convocato per la seconda metà di aprile un Consiglio di Presidenza nel quale la questione sarà affrontata in maniera approfondita, al fine di acquisire gli indirizzi utili ad una definitiva e

nel programmare i concorsi per l'assunzione di personale nella XV legislatura, ha stabilito che entro la fine del quinquennio il numero dei dipendenti dovrà ridursi del 5 per cento rispetto a quello previsto nella pianta organica oggi vigente. Ricordo in proposito che la proposta originariamente formulata dai senatori Questori, nella riunione del 26 ottobre dello scorso anno, al Consiglio di Presidenza, faceva riferimento ad una riduzione nella misura del 5 per cento del personale effettivamente in effettivamente in servizio alla data del 31 dicembre 2006, quindi non alla pianta organica ma al personale effettivamente in servizio. Nel corso di quel dibattito in Consiglio di Presidenza emerse un orientamento conforme al testo attualmente recato dal documento sulle linee guida dell'azione amministrativa che, come è noto, viene proposto al Consiglio di Presidenza e da I senatori Questori - ma credo anche il Consiglio di Presidenza - prendono

assumere questo indirizzo per una serie di considerazioni che qui vi risparmio perché richiederebbero troppo tempo, ma che rinviano certamente ad una valutazione di costi, ad un'azione, che stiamo svolgendo, per procedere al *global service*, al *multiservice* e quindi ad una riduzione di impegno diretto di risorse per avvalersi di maggiori risorse esterne, con

Credo che lo stesso Consiglio di Presidenza, alla luce di questo dibattito e dell'indirizzo da esso emerso, debba tornare a valutare quella determinazione. Concludendo, assicuro che i senatori Questori seguono con attenzione i contatti e i necessari approfondimenti in corso con l'altro ramo del Parlamento in direzione delle possibili interazioni delle strutture di diretto supporto all'attività parlamentare e in particolare a quella di documentazione (Biblioteca, Servizio bilancio e Servizio studi) in modo da conseguire un potenziamento funzionale con risultati di integrazione e di ottimizzazione nell'impiego delle risorse. È stato già ricordato che, per quanto riguarda la Biblioteca, si è già conseguito un risultato. Per quanto riguarda il Servizio del bilancio, siamo determinati nel tener

far maturare delle competenze in sede, in modo tale che le prestazioni di questo nuovo Servizio possano essere da subito disponibili sia per la Camera che per il Senato. Per quanto riguarda gli interventi dei colleghi (mi riferisco ai senatori Grillo, Peterlini, Manzella, De Petris, Santini, Eufemi, Negri, Banti, Galli, Paravia, Ferrara, Manzione, Divina e D'Onofrio) li ringrazio per i significativi spunti di riflessione, di cui i senatori Questori si avvarranno nello svolgimento del proprio mandato e rispetto ai quali ora mi limiterò a brevi considerazioni aggiuntive,

successivamente la nostra valutazione sugli ordini del giorno. In primo luogo, prendo atto - ma l'ho già fatto prima - delle indicazioni di carattere generale sollevate dal senatore Grillo,

Rispondendo ai rilievi del senatore Santini in tema di comunicazione sui lavori del Senato, faccio presente che ai gruppi che visitano il Senato (in particolare le scolaresche, ma anche cittadini comuni) vengono fornite informazioni esaurienti non solo sui palazzi, ma anche sulle modalità dei lavori parlamentari, sul ruolo delle istituzioni, nonché *gadget* e materiale illustrativo. Il Senato, inoltre, è sensibile all'apertura al territorio attraverso la presenza promozionale dello *stand* istituzionale che illustra le funzioni e il ruolo del Senato e la Libreria del Senato, le cui iniziative hanno intensificato, rispetto al recente passato, il rapporto con i cittadini. Per quanto riguarda le richieste di visita dei palazzi, gli uffici del Senato dal giugno 2006 al marzo 2007 hanno ricevuto 1.451 richieste, a seguito sono state fissate per visite guidate e sedute 1.144 appuntamenti. Nell'ambito dei 1.144 appuntamenti, 306 sono stati previsti su richiesta degli onorevoli senatori e 42 su richiesta di onorevoli deputati. Le occasioni in cui i senatori hanno potuto ricevere i gruppi in visita sono state 21 presso la sala delle conferenze stampa che è abbastanza ampia, è adiacente all'ingresso principale di Palazzo Madama

Eufemi, faccio presente che il consuntivo del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori per il periodo 1° gennaio-27 aprile 2006 è riportato alla pagina 31 del corrispondente documento di bilancio. Mi limiterò a sottolineare che la distribuzione dell'avanzo di esercizio

la decisione di tale ripartizione nei due anni successivi contestualmente all'approvazione del rendiconto risponde a esigenze di fluidità nell'azione amministrativa, soprattutto nella prima fase dell'anno finanziario: quando a gennaio o a febbraio non abbiamo ancora avuto la dotazione, abbiamo comunque bisogno di dare continuità all'azione amministrativa e alla spesa degli Uffici. Quanti ai Quanti ai rilievi sulla mancanza di comparazione tra i dati previsti e quelli di consuntivo, questi appaiono ingiustificati alla luce della particolare natura del bilancio di cassa che rende preferibile, in termini di raffronto tra dati omogenei, fare riferimento alle previsioni degli anni messi a confronto. È sempre possibile, naturalmente (se ne terrà conto in futuro), arricchire la significatività indicando anche nei raffronti i dati di consuntivo. Per quello che concerne alcuni rilievi al bilancio del Fondo di previdenza del personale del Senato, che coinvolgono peraltro responsabilità dell'apposito Consiglio di amministrazione di tale istituzione, si ribadisce che il riordino delle prestazioni assicurative garantite dal Fondo è avvenuto senza alcun onere a carico del bilancio del Senato, e non può essere confuso con un contributo di questo tipo l'utilizzo di avanzi che derivano dalla gestione economica del Fondo stesso e che devono essere destinati, per statuto, al miglioramento delle prestazioni per il personale iscritto. Infine, per quanto concerne il collegamento con il sistema informatico SOGEI, si stanno valutando alcuni sistemi di supporto alle decisioni sviluppati dalla predetta società che possano essere utili ai senatori. A tale riguardo sono stati contattati i responsabili delle relazioni esterne di SOGEI e della segreteria del Vice Ministro per avviare un lavoro istruttorio. In relazione a quanto richiesto dal senatore Banti, si comunica che nel corso del 2007 si svolgerà una gara per il rinnovo dei *personal computer* e delle stampanti in uso ai senatori. Tali apparati, che ci auguriamo possano essere disponibili per i senatori all'inizio del 2008, saranno equipaggiati con i più moderni sistemi operativi. Per quanto riguarda l'accenno al Televideo, ricordo ricordo che il Senato, fino alla XIII legislatura, ha utilizzato il servizio, che poi ha dismesso in quanto ritenuto troppo costoso in relazione ai risultati, scegliendo strumenti tecnologicamente più avanzati: sito Internet, *web* TV e canale satellitare. Peraltro, ricordo con piacere che il sito Internet del Senato ha vinto il cosiddetto Nobel in materia: ci eravamo classificati, nell'anno 2005, secondi per tutta la pubblica amministrazione, nell'anno 2006 il Senato è arrivato primo nella competizione tra tutti i servizi di accesso, di conoscenza e di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione. La rassegna stampa estera, infine (è necessario fare una precisazione), non esce una volta alla settimana, ma dal lunedì al venerdì nei periodi di attività parlamentare, ed è un prodotto della Farnesina, da noi riprodotto in una novantina di copie, e fornito *on demand*; quindi, basta chiedere per averla, ove queste novanta copie non fossero sufficienti. La rassegna stampa *on line* del sabato e domenica è molto selezionata e fornita il lunedì, anche in formato cartaceo, così come avviene alla Camera dei deputati. La Camera, peraltro, fornisce una rassegna cartacea più piccola e con uscita ritardata rispetto agli orari del Senato, ed una rassegna *on line* più ricca della nostra. Possiamo farlo anche noi, previa soluzione dei problemi di *storage* che, con gli investimenti che abbiamo realizzato e stiamo completando nel settore dell'informatica, vanno a risolversi. In risposta al senatore Galli, che ha concentrato il suo intervento sulla forte incidenza della spesa per il personale, dirò che certo non voglio eludere il problema, come ho già detto prima, ma quantomeno ricondurlo alle sue esatte dimensioni: infatti il collegio dei senatori Questori, e più in generale il Consiglio di Presidenza, ha ben presente l'esigenza di contenere la dinamica retributiva, e lo stesso bilancio per il 2007 evidenzia questa tendenza; ma devo aggiungere che sia l'aumento registrato nell'arco del 2006, sia quello previsto per il 2007 sono conseguenti ad un accordo sindacale,

che ha portato ad un migliore utilizzo dell'orario di lavoro, ad una maggiore flessibilità nell'utilizzo dell'orario di lavoro, ad un aumento dell'orario di lavoro del personale del Senato e la cui la cui contropartita sono stati anche questi aspetti di carattere salariale. Tuttavia, aggiungo che in termini di valori medi i dati citati nel suo intervento dal senatore Galli non risultano coincidenti con quelli reali, che anzi evidenziano livelli notevolmente più bassi. Ricordo in proposito, come ho già fatto, le valutazioni eccelse sulla qualità, sul rendimento e la professionalità del personale del Senato, unanimemente riconosciute anche all'esterno di questa istituzione e anzi prese spesso a riferimento da altre istituzioni della Repubblica. Con riguardo all'intervento del senatore Ferrara, posso in primo luogo comunicare che, anche a seguito di studi condotti nel passato sull'informatizzazione dell'Aula del Senato e delle Aule di Commissione, nei prossimi mesi, sulla base dello stato di avanzamento del piano di realizzazione della nuova rete informatica, il Collegio dei Questori esaminerà un piano di diffusione nei palazzi del Senato della tecnologia *Wi-Fi*. Per quanto riguarda l'intervento del senatore Manzione, debbo intanto informare che sono in corso contatti, speriamo, risolutivi tra i Gruppi parlamentari per la definitiva attuazione del posto fisso in Aula, tenendo conto che la parte informatica e strutturale, di competenza del Collegio dei Questori, è stata da tempo realizzata e collaudata, cioè che quest'Aula è pronta per poter utilizzare il posto fisso in Aula.

alla senatrice De Petris. L'ordine del giorno G1 è accolto come raccomandazione, in quanto le istanze contenute sono pienamente condivise e, in ogni caso, sono parte non secondaria della più generale politica di risparmio voluta con determinazione dai senatori, come si evince dal consuntivo 2006, con

Nella valutazione della spesa relativa alle risorse energetiche non va, in ogni caso, trascurata la circostanza dei notevolissimi aumenti registrati nel comparto in questi ultimi anni, che si riflettono ovviamente sugli andamenti della spesa del nostro bilancio. Dal punto di vista dei costi, sono già stati razionalizzati i contratti con ACEA e Italgas, con positivi effetti di risparmio che dovrebbero già registrarsi a partire dall'esercizio in corso. Occorre pertanto proseguire in tale direzione per ottenere ulteriori economie. Quanto alla lievitazione delle spese energetiche, l'incremento in linea generale è legato all'andamento delle tariffe. Il *trend* anomalo, in termini di cassa, sul bilancio 2004 è piuttosto l'effetto di trascinamento dovuto a ritardate fatturazioni, per cui le spese di competenza di un esercizio possono risultare effettivamente liquidate in quello successivo o addirittura due anni dopo. Il Collegio chiede sin d'ora all'Amministrazione di impegnarsi nel contenimento dei consumi energetici attraverso le seguenti iniziative: la centralizzazione, ove possibile, dei servizi energetici (riscaldamento, rinfrescamento e acqua calda sanitaria), che consente un'economia di scala rispetto alle singole produzioni locali; il controllo del fattore di potenza dell'energia elettrica su tutti i circuiti alimentati; ove possibile, il ricorso alle lampade fluorescenti in sostituzione di altri sistemi di illuminazione più energivori; il ricorso a materiali non solo impiantistici con alto coefficiente termico, che consenta il contenimento delle dispersioni termiche; la revisione dei parametri di temperatura ambientale utilizzati dai sistemi di climatizzazione caldo-freddo verso più basse temperature d'inverno e più alte d'estate, naturalmente con il consenso di tutti gli utenti. Viene quindi accolto l'indirizzo fornitodai presentatori dell'ordine del giorno nel senso di aumentare l'efficienza energetica delle strutture del Senato. Riteniamo che la specifica qualificazione di alcune competenze professionali presenti presso le strutture amministrative dell'Amministrazione siano sufficiente

e le competenze relative con il personale già a disposizione. Quanto all'ordine del giorno G2, per l'utilizzo di materiali pericolosi o a significativo impatto ambientale, l'Amministrazione sta provvedendo già da qualche anno alla loro eliminazione e sostituzione con altri materiali nel rispetto delle normative vigenti. In particolare, tale attività di eliminazione e sostituzione, svolta nel recente passato, viene effettuata sistematicamente in occasione di ristrutturazioni o interventi di manutenzione edile ed impiantistica. Per quanto riguarda lo smaltimento differenziato dei rifiuti, la quasi totalità dei rifiuti costituita da carta viene donata alla Croce Rossa attraverso un intermediario. Ricordo che il resto dei rifiuti viene differenziato prima dello smistamento, dividendolo in ben 11 diverse categorie, che vi risparmio. L'ordine del giorno pertanto può essere accolto come raccomandazione, ricordando infine che la dimensione dell'utilizzo di carta va in riduzione con il diffondersi e l'implementarsi del sistema informatico che ha come effetto...

risolvere non solo da noi, che lo avevamo già fatto nella scorsa legislatura, ma dalle due più alte cariche di Camera e Senato, quindi dal presidente Bertinotti e dal presidente Marini. La Camera ha pensato di affrontare la questione in un determinato modo. Il presidente Marini, credo più opportunamente, ha deciso di affrontarla in modo più strutturale nel senso che è stata istituita una Commissione presieduta dal Presidente della Commissione lavoro che riordinerà il sistema delle norme di lavoro esistenti al riguardo, eventualmente innovandole pervenire ad una soluzione definitiva e strutturale della materia. Per quanto riguarda le considerazioni svolte dall'ordine del giorno G5 del senatore Manzione, sono certamente interessanti e meritevoli di approfondimento perché aprono una riflessione che è in linea con i tempi e con i ragionamenti che abbiamo fatto finora parlando dei costi della politica in generale. Infine, i chiarimenti al presidente D'Onofrio sull'assegno vitalizio di reversibilità: nessun diritto per il convivente. Può essere liquidato al coniuge finché resta nello stato vedovile; ai figli minorenni; a quelli maggiorenni se inabili a proficuo lavoro; in assenza di altri titolari, a genitori o fratelli nullatenenti e a carico. Quindi il chiarimento che lei ha chiesto è già stato fornito da lei medesimo. Non si tratta da parte nostra che di ribadire quanto da lei affermato. all'assegno di fine mandato, in caso di premorienza del senatore a carico si indica un qualunque beneficiario, persone fisiche o giuridiche (possono cioè essere anche enti, e così via). Questo vale

quanto riguarda l'assistenza sanitaria, il titolare può iscrivere il convivente *more uxorio* dopo tre anni di convivenza o se ci sono figli

ringrazio, senatore Nieddu: lei di tutto potrà essere accusato meno che di evasività, stia tranquillo, di questo non la accuserà mai nessuno.

nemmeno non avere l'attenzione di contrastare una deriva antipolitica che di qualche precisazione ha bisogno; questo cercheremo di farlo.

ora agli ordini del giorno,

di mandati non superiore a due: anche quello è un modo ovviamente per porre la questione. Questo tenevo a dirlo; credo che questo sia lo spirito con cui noi abbiamo lavorato.

per supportare il lavoro parlamentare e l'attività legislativa. Perché questa (lo richiamava anche il senatore Manzella nel lavoro sulle Commissioni) è la

Presidente, noi esprimiamo un voto favorevole al bilancio e lo facciamo per una serie di motivazioni che rapidamente cercherò di evidenziare. Prima però vorrei fare una riflessione di ordine generale: noi affrontiamo il dibattito sul bilancio interno del Senato e mai, come in questo caso,

relatore, sulla centralità del tema del costo della politica e del ruolo, della funzione, della politica. Se mi è consentita una battuta, parliamo tanto di questioni previdenziali, ma uno dei pensionamenti che dobbiamo evitare è il prepensionamento della politica, perché il rischio è che la politica, il suo ruolo, la sua funzione ineliminabile, si dissolva, si disperda, perdendo di ruolo, significato e funzione. significato e funzione. Queste valutazioni danno al dibattito che abbiamo svolto e stiamo svolgendo un'accentuazione importante e significativa, per cui è responsabile e doverosa l'attenzione su alcune questioni, ancora di più rispetto a prima. La prima questione è esattamente quella del personale. Credo siano stati fatti dei passi in avanti importanti e ritengo che l'approvazione del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità del giugno 2006 sia stato un fatto rilevante e significativo. Non basta. Bisogna continuare in questa opera di modernizzazione molto forte e significativa. Il senatore Eufemi faceva prima riferimento al controllo di gestione, cioè al tema del bilancio di cassa e del bilancio di competenza. Ci sono varie questioni che vanno ulteriormente affrontate

la questione previdenziale relativa al personale assunto dopo il 1998. C'è un tema ulteriore che riguarda il personale e che dobbiamo affrontare e approfondire:

per le norme approvate dal Parlamento, debbono far riferimento alla dotazione organica riferita al 31 dicembre 2006. È vera anche la la riflessione, fatta dal collega Nieddu, rispetto all'*iter* che questa vicenda ha avuto nel dibattito all'interno del Consiglio di Presidenza. È giusto che si prenda atto di quello che è emerso ed è giusto che su questo ci sia un approfondimento che porti a definire il rapporto con la dotazione organica, eliminando quel riferimento alla pianta organica che oggettivamente si presta, proprio rispetto alle riflessioni iniziali, ad una chiara valutazione equivoca (che è preferibile evitare, proprio per dare il massimo del rigore e della serietà all'impostazione che tutti siamo interessati a seguire in questa fase).

il massimo della qualità e del merito per cercare di rispondere nel modo migliore all'esigenza che è stata prospettata e che ci richiamerebbe però ad una riflessione - il presidente Morando lo sa meglio di me - un po' più ampia riguardante riguardante un riassetto complessivo istituzionale rispetto alla vicenda. Non è ad ogni modo questa la sede per affrontare la questione; questo è uno spicchio di un problema ben più ampio e significativo. Per il resto, credo sia utile accelerare notevolmente sul versante di una modernizzazione sia rispetto ai servizi, sia rispetto alle esternalizzazioni (il tema, che è stato affrontato, del *global* *service* e del *multiservice***;** mi limito soltanto al titolo, più che al merito della questione)

che sottolineano alcuni elementi di positività ma intravedono anche ulteriori elementi di criticità e alcuni nodi che inevitabilmente bisognerà sciogliere, con questa impostazione processuale

Signor Presidente, visto che sono stati dati i numeri dell'*audience* mi fa piacere sottolineare che, per ascoltare la replica del Collegio dei senatori Questori, l'Aula si sia un po' riempita. Significa che c'è quella giusta attenzione per questo importante strumento dell'approvazione del bilancio del Senato. Vorrei dire un grazie al Collegio dei Questori, al senatore Nieddu in particolare, alla collega Thaler Ausserhofer e al collega Comincioli, ma anche a tutto il Consiglio di Presidenza. In effetti, in questo primo anno di esperienza credo che siano stati conseguiti buoni risultati. Uno è stato segnalato da tanti colleghi: il fatto che finalmente abbiamo recuperato l'anno di ritardo che avevamo sulla presentazione dei rendiconti. Questo è molto importante, perché finalmente siamo in condizione di capire, con una certa trasparenza, che cosa avviene nei conti pubblici del Senato, e quindi è sicuramente un fatto positivo. segnalo che è molto positivo che discutiamo e approviamo il bilancio preventivo praticamente all'inizio di aprile, quando normalmente, nella vita del Parlamento, di tutti e due i rami

si misura sui risultati. Ovviamente non si è fatto tutto - tra poco ascolteremo il collega Manzione -, ci sono ancora delle delle lacune, però sento di poter dire che il servizio che ha reso il Collegio dei Questori è sicuramente positivo.

che mette tutti i senatori in condizione di avere una presenza più tranquillizzante, più serena e servizi migliori per tutte le necessità. Ma il mio plauso è, più in generale, per il rigore

vorrei che fosse chiaro che, rispetto ai 503 milioni di euro previsti nel triennio, nel 2006 noi abbiamo speso 14 milioni in meno.

i Questori ci propongono di votare un bilancio che prevede di spenderne 503, con un risparmio di 23 milioni di euro.

per il 2006 è stata di 14 milioni in meno, per il 2007 sarà di 26 milioni in meno ed è previsto che per l'anno prossimo sarà

i colleghi assenteisti (che ci sono, come in ogni famiglia), cioè quelli che non sempre frequentano i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni, ma sarebbe opportuno che il Consiglio di Presidenza adottasse un regolamento per le trattenute

noi non funzioniamo al *top* perché il rapporto Commissioni-Aula è sfasato: non può essere che il momento di elaborazione effettiva della legge,

per avviare il processo di federalismo istituzionale attraverso la partecipazione delle Regioni ai lavori delle Commissioni che si occupano dei problemi regionali. È stato svolto un lavoro preparatorio nella scorsa legislatura ed io credo che si debba dare avvio a tale processo e si debba anzi regolamentare la partecipazione delle Regioni alla vita del Senato proprio perché ciò favorirebbe quel processo di federalismo istituzionale da tutti auspicato. In ultimo, non perché è un dovere ma perché lo sento, voglio rivolgere un ringraziamento al Segretario Generale, a tutti i dipendenti del Senato ed in particolar modo a quelli ai quali do più noia, gli amici del Servizio dell'Assemblea; penso che tutti i colleghi senatori siano molto soddisfatti dei servizi che essi rendono a noi ed indirettamente al Paese.

relativi agli aspetti previdenziali e all'accesso alle cariche elettive; egli ha pronunciato parole chiare anche rispetto ad un passato lontano degli eletti per censo, delle quali lo ringrazio.

era quanto volevamo e quindi il chiarimento è stato opportuno. Bene ha fatto il presidente Marini a respingere attacchi strumentali di antiparlamentarismo che vanno contrastati con un'efficace comunicazione. interno oggi in esame assume un fortissimo significato sia per il livello della spesa che per le scelte sottostanti. Forse hanno prevalso ragionamenti più sull'azienda Senato che non sulla istituzione Senato. Da parte nostra restano preoccupazioni in ordine a questioni che rischiano di riverberarsi sul funzionamento dell'istituzione. Riteniamo che la parte più rilevante sia la questione relativa alle risorse umane, che dobbiamo salvaguardare nel più alto livello. Esprimiamo, quindi, apprezzamento per il lavoro che quotidianamente svolgono, dal Segretario generale all'ultimo dipendente, in termini di autonomia, formazione, competenze e professionalità. Tutto ciò è più efficace ed importante quanto più ci si muove all'interno di una cornice di regole che fanno parte della storia delle istituzioni, della consuetudine delle istituzioni e dell'affermazione di un principio, che è quello della separazione tra politica e *management*, senza invasioni di campo.

dei compiti, perché avvicina i cittadini alle istituzioni ed accresce il dialogo tra elettori ed eletti. Il nostro auspicio è che prevalga in questo progetto di bilancio, insieme ai documenti contabili, contabili, un uso razionale delle risorse, perché dall'efficienza, dalla modernizzazione e dalla funzionalità del Senato deriva il rafforzamento delle istituzioni del Paese. Il mio intende essere soltanto uno stimolo costruttivo a lavorare meglio, valorizzando le risorse umane di cui siamo dotati, perché valorizzare l'istituzione Senato significa rafforzare la democrazia del Paese.

anche ringraziare il Collegio dei Questori per le risposte che ha fornito su alcuni temi da me proposti, relativi, ad esempio, alle visite e alle problematiche che ho segnalato. Ho preso atto dei numeri dei visitatori e dei gruppi che sono entrati; non c'è, purtroppo, la controprova, senatore Nieddu, di tutti i gruppi che si sono sentiti non era possibile entrare perché era necessario un anno di attesa. Il mio è un voto di buona volontà. Vi prego di verificare se esistano le condizioni per migliorare questo *trend*, per accorciare i tempi di attesa. Molti hanno toccato un tema che forse è solo indirettamente collegato al bilancio del Senato: la nostra condizione di indennità e soprattutto di vitalizio. Ho lanciato quella che poteva sembrare una provocazione ma che è, viceversa, una mia profonda convinzione; nessuno l'ha raccolta, né per negarla né per criticarla, né, tanto meno, per dichiararsi d'accordo. Ho proposto che il cittadino che venga eletto ad una carica parlamentare non abbia un'indennità in più rispetto allo stipendio di cui già gode come lavoratore, ma trasferisca nella sua nuova condizione di parlamentare il proprio livello salariale, la propria anzianità e soprattutto il proprio trattamento previdenziale (in modo da escludere una indennità di carica, un secondo stipendio), maturando per scatti di anzianità o con le dinamiche che la sua categoria prevede quei miglioramenti che avrebbe rimanendo sul proprio posto di lavoro.

di fronte ai cittadini che mi dicono che il vitalizio è un privilegio. Cerchiamo di renderci conto che fuori di qui non sono tutti ciechi e sordi. Caro senatore Nieddu, lei ha giustamente

3.100 euro dopo cinque anni, francamente, nessuna categoria li prevede. Il fatto che - come ha ricordato lei - anche i parlamentari europei e i consiglieri regionali

la lettura che ho svolto di quelli tenuti in passato: debbo rilevare che, se oggi si sono raggiunti risultati da parte del Collegio dei Questori, è perché si è partiti da lontano nel cercare di introdurre temi di responsabilità,

centrano l'obiettivo di un bilancio che registri e contemperi la necessità di trasparenza e di rigore con quella di salvaguardare non già i privilegi, ma le prerogative. Non vorrei che questo si appuntasse

(così come, in alcuni casi, non apprezzo quanto sostiene anche in altre sedi). Perché non l'ho fatto? Perché, con l'intervento e con gli ordini del giorno, erano stati posti quattro temi.

la previdenza dei dipendenti, rispetto alla quale avevamo proposto un modello (una soluzione di modello o un modello per la soluzione) e non una soluzione di merito, al di là delle parole in questo caso pronunciate, interessante e meritevole. Non mi pare vi sia stata una valutazione concreta nel merito nel merito di quella vicenda, che, però, andrebbe approfondito, per non dare una risposta, come sempre, assolutamente insoddisfacente. Avevo chiesto, con l'ordine del giorno G4, firmato anche dal collega Calvi, di garantire la necessità di fare in modo che la terzietà e l'indipendenza degli organi di autodichia venisse rispettata: non c'è stata nessuna risposta, così come per l'impegno dell'indicazione nella spesa delle risorse per le spese di rappresentanza. Ecco perché, per la simpatia che nutro per il collega Boccia, dal quale mi devo purtroppo dissociare, e per la stima per la Presidenza, trasformo la mia contrarietà in un voto di mera astensione.

la dovuta energia una presa di distanza da questa canea di una campagna di stampa populista e neopauperista, da parte anche di giornalisti che mediamente, per scrivere sessanta righe al giorno, quando le scrivono, guadagnano dagli 8.000 ai 10.000 euro al mese; mi riferisco ai giornalisti dei quotidiani «Corriere della sera», «La Stampa», «la Repubblica», anche perché provengo da quella categoria e so bene quanto guadagnano e quanto parassitismo alligna nei giornali. Credo che un ceto politico, una classe dirigente che si vergogna del proprio *status* e che si fa travolgere da queste campagne pauperistiche e populistiche non sia degna di rivestire il ruolo che pretende di rivestire. In realtà, in questo Paese c'è gente, anche nel pubblico impiego, che può accreditarsi appannaggi molto più consistenti di quelli parlamentari,

tutto è superfluo). Però un parlamentare, e soprattutto un parlamentare del Mezzogiorno, deve fare i conti con una richiesta di presenza politica articolata e che punta, a volte, a risolvere anche problemi che dovrebbe risolvere lo Stato sociale e che lo Stato sociale non è in grado di affrontare. Allora

una sottolineatura di quanto gli atti ispettivi non si limitino soltanto a prospettare argomenti di interesse parlamentare, ma ma puntino a volte a prevenire i problemi che possono derivare dall'inerzia del Governo e di organi dello Stato. Ho sollecitato quattro volte questa interpellanza, presentata il 7 febbraio, a proposito della detenzione di Mario Scaramella;

preventivo senza evidentemente alcuna condanna, è stato ricoverato in ospedale ed è in condizioni davvero gravi. Ritengo che più che mai sarebbe dovere del Ministro venire a rispondere con urgenza. Sarebbe dovere del Ministro dar segno di interessarsi a questa vicenda, che pure ha sollecitato quando, prospettandosi il rientro in Italia di Mario Scaramella e di conseguenza il suo arresto (poiché Scaramella sapeva che lo aspettava l'arresto e nonostante questo è tornato in Italia), si è augurato che le

senza che alcunché sia emerso. Anzi, studiando il caso emerge che nell'anno e due mesi durante i quali la fonte segnalata da Scaramella quale provenienza delle accuse da lui formulate nei confronti di alcuni cittadini ucraini, arrestati perché trovati in possesso dei sistemi d'arma da lui

di una persona che, arrestata da tre giorni, ha tentato il suicidio, credo dovrebbe avere la sensibilità di interessarsi anche della salute di Mario Scaramella, nonché dell'interpellanza da me presentata il 7 febbraio scorso. Senatore Malan, le posso rispondere che l'impegno è quello che abbiamo già fissato: una riunione apposita del Senato per discutere le interrogazioni e le interpellanze che riguardano la giustizia, nella quale faremo in modo che

Si era riusciti a farle avere il permesso per essere curata presso l'ospedale San Carlo di Potenza, dove era ricoverata da circa un anno,

l'intervento di trapianto era anche stato predisposto e concordato con il Policlinico Umberto I di Roma. Ebbene, la ragazza ieri è deceduta.